L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Con la conversione del decreto-legge n. 113 del 2016, recante misure urgenti per gli enti territoriali, è stato risolto il problema delle cosiddette precarie degli asili nido da oltre trentasei che rischiavano il mancato rinnovo del contratto. La norma, fortemente sostenuta dal Governo, consente il regolare avvio dell'anno scolastico. Essa, infatti, consente ai Comuni di procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa. Ciò garantirà la continuità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, come già avviene per il sistema nazionale di istruzione e formazione, e verrà così assicurata la qualità del servizio medesimo. Inoltre, per non disperdere le professionalità acquisite dal suddetto personale impegnato con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai Comuni è consentito di procedere all'assunzione di personale presente in graduatoria, nonché del personale che verrà inserito in altre graduatorie da definirsi a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Sono state autorizzate procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, con tre anni di servizio, anche non continuativi, a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento. Il Governo, dunque, con un intervento straordinario, ha dotato gli enti locali di ogni utile strumento per risolvere un problema di elevata sensibilità sociale, consentendo - come anche richiesto dall'interrogante - di superare anche il limite del *turnover*, previsto per il 25 per cento, delle cessazioni. Adesso spetta ai Comuni utilizzare al meglio questi strumenti, non vanificando lo sforzo che ha dato vita a questo impegno eccezionale. Tra le città che avevano segnalato il problema e che avevano dimostrato di avere effettive difficoltà a iniziare l'anno scolastico, segnaliamo che alcune di esse hanno già attivato abbondantemente le produrre - mi riferisco alle città di Torino. Bologna, Milano, Genova e Rimini - mentre altre hanno iniziato ma fanno più fatica. Penso al Comune di Roma, che aveva segnalato particolare difficoltà di scoperto in organico e di contratti che andavano in scadenza. Ci auguriamo, quindi, che tutte le amministrazioni

avrebbero avuto diritto di vedere finalmente riconosciuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; al livello nazionale paradossalmente questo stava accedendo e invece vi erano molti impedimenti a livello locale. Lei però tra tutti i Comuni non ha indicato il Comune di Roma,

per un posto di coadiutore amministrativo presso il Dipartimento prevenzione veterinaria della ASL di Pavia. L'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attribuisce all'Ispettorato per la funzione pubblica

delle sue funzioni ed al fine di assicurare il rispetto del principio del merito, richiamato da ultimo dall'articolo 17 della legge n. 124 del 2015, l'Ispettorato, su impulso del Ministro, ha avviato un'attività di indagine per comprendere le motivazioni che hanno portato all'annullamento della procedura concorsuale cui si riferisce l'interrogante. Il direttore generale della ASL di Pavia, facendo seguito alla richiesta dell'Ispettorato, con nota avente numero di protocollo 43415/2016 del 29 luglio 2016, ha precisato che la procedura di reclutamento avviata non riveste i caratteri di concorso pubblico, in quanto non è stato pubblicato alcun formale bando sulla *Gazzetta Ufficiale* e non è stata costituita un'apposita commissione d'esame con la presenza di componenti esterni all'ente. La ASL ha quindi sostenuto che si tratta di prove attitudinali volte alla sola valutazione di idoneità. La ASL però, prima di dare corso a questa procedura, ha richiesto al centro per l'impiego di Pavia di fornire la graduatoria dei nominativi che avessero i requisiti idonei per la posizione richiesta. Delle 64 persone iscritte nella suddetta graduatoria, solo 47 hanno partecipato alla selezione; la prima ed unica idonea al posto da ricoprire è stata la signora Daniela Cosentino, che aveva già avuto precedenti esperienze lavorative all'interno dello stesso Dipartimento, con contratti di lavoro a tempo determinato ed atipici. Nell'analizzare il lavoro della commissione, la ASL ha constatato che la stessa non si è limitata esclusivamente ad una valutazione di idoneità, ma ha utilizzato criteri, sia per la definizione delle domande che per la valutazione delle singole prove, oltrepassando, a giudizio dello stesso ente che aveva avviato la procedura, i criteri posti alla base della selezione. Conseguentemente, la ASL ha deciso di agire in autotutela e con il decreto n. l37 del direttore generale del 12 luglio 2016, 2016, chiarendo i motivi di annullamento della selezione, senza tuttavia annullare *in toto* le precedenti fasi in base al principio della conservazione degli atti amministrativi, dando così la possibilità a tutti i partecipanti - i che avevano risposto positivamente - di effettuare nuovamente le prove. Alla luce di quanto esposto dalla ASL, l'Ispettorato per la funzione pubblica ha richiesto ulteriori specifiche all'amministrazione interessata, interessata, ritenendo che oggi non risultino evidenti le motivazioni a supporto dell'azione amministrativa che è stata seguita dall'ente. Quindi, a fronte di questa ulteriore osservazione, l'ispettorato ha chiesto ulteriori chiarimenti e specificazioni tenendo ben presente che ci troviamo all'interno di una competenza esclusiva in materia sanitaria della Regione e che, quindi, l'ASL quindi, l'ASL è sottoposta a poteri di controllo, vigilanza e indirizzo da parte della Regione stessa e che il Governo, da questo punto di vista, non ha poteri sostitutivi nei confronti della Regione per poter attivare procedure diverse.

lesioni di diritti nei confronti dei partecipanti o della persona che sia risultata idonea o se, invece, come ritiene la ASL, siano state rispettate tutte le regole ad oggi vigenti. [DI

Signor Presidente, con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, riguardante lo scarico nel sottosuolo delle acque derivanti dall'estrazione e dalla separazione di idrocarburi del Centro Olio Val d'Agri di Viggiano, sulla base degli elementi acquisiti da apposita direzione generale, nonché dagli enti nazionali e territoriali competenti, si rappresenta quanto segue. L'ENI, a seguito del sequestro preventivo da parte dell'autorità giudiziaria di alcuni impianti del Centro Olio Val D'Agri (vasche asservite all'unità 560 e pozzo di reiniezione «Costa Molina 2»), lo scorso mese di aprile ha reso noto di aver proceduto alla chiusura graduale della produzione dei pozzi, nonché alla fermata generale temporanea degli impianti del Centro Olio Val D'Agri. La Regione Basilicata, con la delibera di Giunta del 12 aprile 2016, ha disposto la sospensione dell'esercizio dell'attività di scarico in unità geologiche profonde delle acque di strato mediante il pozzo «Costa Molina 2» con effetto immediato e per un periodo non superiore a novanta giorni, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento.

A seguito della conferma del sequestro sentenziata dal tribunale del riesame di Potenza il successivo 16 aprile, L'ENI ha avviato un programma di messa in sicurezza e conservazione dell'*asset* del Centro Olio Val d'Agri e dei pozzi ad esso afferenti della durata di sei mesi, che include tutte le attività e interventi da realizzare sulle tre macroaree: rete di raccolta, Centro Olio Val d'Agri, oleodotto COVA-Taranto. Di questo programma di interventi la stessa ENI ha informato la Regione e l'ARPA Basilicata. L'autorità giudiziaria in data 1° giugno 2016 ha disposto il dissequestro temporaneo delle due vasche e del pozzo di reiniezione Costa Molina 2 al solo fine di consentire la realizzazione delle opere e dei lavori indicati negli atti, così come disposto dai pubblici ministeri, stabilendo come termine ultimo il 31 agosto 2016 per la loro realizzazione, ovvero anche prima di tale data, qualora la società dovesse dichiarare l'avvenuta ultimazione delle opere di adeguamento. Nello stesso mese di giugno, l'ENI ha comunicato alla Regione Basilicata la richiesta di «modifica non sostanziale» dell'impianto per l'attuazione di interventi finalizzati all'adeguamento dell'impianto agli elementi tecnici avanzati dall'autorità giudiziaria connessi alla gestione delle acque di strato prodotte durante l'esercizio del Centro Olio Val d'Agri. Con apposita delibera di Giunta regionale del 25 luglio è stata autorizzata la ripresa dell'attività del pozzo Costa Molina 2 e, in data 4 agosto, la procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza ha espresso parere favorevole al dissequestro delle vasche e del pozzo Costa Molina 2. Per quanto attiene alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, nel maggio scorso l'ARPAB ha fornito i dati relativi alle indagini analitiche effettuate sulle acque sotterranee dell'area limitrofa al pozzo di reiniezione Costa Molina 2 tra il gennaio 2014 e l'ottobre 2015. Tali analisi, effettuate su campioni di acque prelevati dalle sorgenti denominate SG4 e SG8, hanno fornito nel periodo indicato valori sempre inferiori al limite di rilevabilità analitica. Sempre l'ARPAB ha integrato ulteriormente la documentazione con gli esiti analitici relativi alle acque superficiali dell'invaso del Pertusillo, destinate alla produzione di acqua potabile, di cui all'articolo 80 del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tali analisi, condotte negli anni 2014 e 2015, evidenziano che, nel punto specifico di campionamento dell'invaso del Pertusillo situato in prossimità del punto di captazione delle acque ad uso potabile, gli idrocarburi, sia totali che aromatici, sono risultati inferiori rispetto ai valori parametrici previsti dal citato decreto legislativo. Per quanto attiene al rischio legato all'attività sismica dell'area, si precisa che il Ministero dello sviluppo economico ha elaborato delle linee guida per le attività minerarie quali estrazioni e reiniezione di fluidi, da applicare per il monitoraggio e la prevenzione del rischio sismico. Il documento è stato redatto anche in collaborazione con sismologi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e di altre istituzioni di ricerca. Le indicazioni contenute nelle linee guida prevedono che le reiniezioni devono essere effettuate solo con pressioni di fluidi

dall'altro le analisi fatte da privati ci dimostrano esattamente il contrario. Abbiamo situazioni sia di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), sia di materie pesanti che sono presenti in un bacino idrico. Ricordiamo che il pozzo Costa Molino 2 è vicino al lago del Pertusillo, un bacino d'acqua potabile che dovrebbe fornire acqua finanche in Puglia. Purtroppo la situazione rimane nella sua totale gravità. Chiediamo che il Governo faccia quanto è nelle sue possibilità e di fare pressione sull'ARPA in modo tale che ci sia un continuo monitoraggio, perché non è possibile che le analisi di cui parliamo risalgano al 2014-2015. Dovremmo effettuare un monitoraggio continuo affinché si capisca almeno da dove vengono questi inquinanti, che - ripeto - ci sono, esistono e, purtroppo, stanno mettendo la Basilicata in una condizione in cui la gente si ammala e muore.

con riferimento all'interrogazione relativa al fenomeno dei roghi di rifiuti in Campania, sulla base degli elementi acquisiti dall'apposita direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle altre amministrazioni competenti, si rappresenta quanto segue. Secondo quanto riferito dall'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione Campania, presso la prefettura ufficio territoriale di Napoli, l'andamento del fenomeno dei roghi di rifiuti è costantemente monitorato dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco di Napoli e di Caserta. A partire dal 2013 - anno in cui sono state potenziate le attività di contrasto e prevenzione del fenomeno - gli interventi di spegnimento di incendi di rifiuti da parte dei Vigili del fuoco evidenziano un *trend* in netta diminuzione. I dati relativi al 2015 confermano ed ampliano la tendenza in calo, con meno del 63 per cento in Provincia di Caserta e meno del 42 per cento in Provincia di Napoli. Gli incendi sono ascrivibili a condotte e cause disomogenee. Una parte è conseguenza di pratiche di smaltimento abusivo dei rifiuti, anche speciali; alcuni incendi avvengono in prossimità dei campi rom, in aree utilizzate abusivamente per il deposito e lo smercio di materiali; il maggior numero degli interventi dei Vigili del fuoco si concentra, infine, nel territorio urbano di Napoli. La riduzione degli interventi di spegnimento ha riguardato in questi anni tutte le tipologie di incendio e ogni tipo di materiale, in particolare quelli più pericolosi, come confermano le statistiche relative ai primi mesi dell'anno in corso: da gennaio ad aprile non si è verificato infatti in Provincia di Caserta nessun incendio di pneumatici, mentre nella Provincia di Napoli sono stati otto contro i 39 dei primi quattro mesi del 2012. I risultati ottenuti sono frutto dell'impegno con il quale le istituzioni, le Forze dell'ordine, l'Esercito, gli enti locali, le associazioni ambientaliste e i comitati civici aderiscono alle attività promosse nel quadro del patto per la terra dei fuochi, stipulato su iniziativa dell'incaricato del Governo per il fenomeno dei roghi di rifiuti in Campania e coordinate dallo stesso presso la cabina di regia interistituzionale con le prefetture, la Regione Campania e gli enti locali. Tra le numerose misure adottate si evidenziano, in particolare, quelle dedicate al potenziamento dei controlli delle Forze dell'ordine, che si avvalgono anche del concorso straordinario di 200 militari dell'Esercito, assegnati ai prefetti di Napoli e di Caserta. Allo scopo di rendere più incisiva la repressione, è stato peraltro istituito, presso l'ufficio dell'incaricato del Governo, un tavolo di lavoro con le procure, le Forze dell'ordine e le

che ha introdotto i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale ed omessa bonifica, avviando, d'intesa, una specifica attività di formazione interforze per *detective* ambientali, che ha coinvolto oltre 300 uomini delle forze di polizia, dei Vigili del fuoco, delle polizie locali. In parallelo, sul piano amministrativo, sono in corso misure per il supporto giuridico, tecnico e finanziario in favore dei novanta Comuni aderenti al favorendo interventi di bonifica, riqualificazione e telecontrollo del territorio, e il prelievo gratuito degli pneumatici abbandonati con oltre 10.000 tonnellate di gomme recuperate e sottratte ai roghi. Per ampliare il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste e civiche è stata attivata, tra l'incaricato del Governo e la Federazione delle associazioni e dei comitati civici, in attuazione del programma «Europa per i cittadini», la rete degli osservatori civici per la tutela della salute e dell'ambiente, con oltre 500 aderenti. L'attivazione e la partecipazione della cittadinanza si avvale inoltre dell'applicazione per *smartphone* «Aiutaci a spegnere i fuochi», che consente ad ogni cittadino di attivare gli interventi dei Vigili del fuoco, dei Comuni e delle Forze dell'ordine sui luoghi di incendio e di abbandono dei rifiuti.

Tale documento è attualmente in corso di istruttoria. La sua approvazione, fermi restando gli aspetti di natura finanziaria, consentirebbe di rafforzare ulteriormente l'attività di prevenzione e di contrasto al fenomeno dello smaltimento abusivo e dei roghi, essendo previsto il consolidamento e l'ampliamento delle azioni in corso e l'attivazione di nuove linee operative. Per quanto concerne, infine, l'articolo di stampa citato dal senatore interrogante, esso si riferisce agli incendi avvenuti a cavallo dei mesi di giugno e luglio dello scorso anno a Giugliano, in prossimità delle aree vaste ex SIN, e comprendente una serie di siti di discarica, tuttora oggetto di sequestro giudiziario. Su tali aree sono state effettuate indagini e sono in corso interventi di messa in sicurezza, a cura del commissario delegato. Gli episodi incendiari, sui quali procede il tribunale di Napoli Nord, non sono imputabili ad un'unica matrice. In seguito agli stessi, sono stati ulteriormente rafforzati a Giugliano i servizi di vigilanza ravvicinata nei pressi delle aree interessate maggiormente dagli incendi; sono stati intensificati i servizi di polizia lungo le strade di collegamento verso i siti di stoccaggio abusivo dei rifiuti e nelle aree di illegale sversamento, finalizzati all'individuazione dei responsabili nonché al sequestro dei mezzi impiegati per il trasporto del materiale. Sono stati, altresì, ulteriormente potenziati i controlli sulle attività economico-produttive per la verifica delle procedure di smaltimento dei rifiuti e del materiale di scarto. A ciò si aggiungono gli interventi effettuati nell'ambito del Patto per la Terra dei fuochi, che hanno consentito di recuperare circa 1.500 metri cubi di rifiuti - urbani e speciali - in luoghi, da decenni interessati da pratiche di scarico abusivo, dei quali è prevista anche la riqualificazione con la dotazione di telecamere, collegate con le sale operative della polizia locale e delle Forze dell'ordine. A seguito di queste attività, i roghi nel territorio di Giugliano sono stati drasticamente ridotti. Per completezza di informazione si fa presente inoltre che, secondo quanto riferito dall'ARPA Campania, la stessa ha previsto, nell'ambito delle attività disciplinate dalla legge n. 6 del 2014, di indagare numerosi terreni agricoli ricadenti nell'intera area vasta di Giugliano, per individuare quelli non idonei alle produzioni agricole, per la presenza di contaminanti legati proprio agli incendi e allo smaltimento illegale dei rifiuti. In questo contesto, negli ultimi due anni, numerosi terreni e colture agrarie del comprensorio in questione sono stati già indagati e i risultati sono pubblicati sul sito *web* dell'Agenzia, dove è possibile osservare anche la localizzazione dei terreni investigati, che risultano limitrofi alle discariche più attenzionate. Tali indagini si aggiungono a quelle copiose che ARPAC ha già effettuato negli anni precedenti su richiesta del Commissario di Governo delegato nell'ambito delle attività di propria pertinenza, inerenti la messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e dei laghetti di Castelvolturno. Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, il Ministero dell'ambiente prosegue nella sua azione costante di monitoraggio senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tali tematiche, anche al fine di valutare eventuali coinvolgimenti di altri soggetti istituzionali.

È vero, sì, che a Giugliano in parte il problema è stato risolto, ma si è spostato verso Casal di Principe e, in parte, nella provincia di Napoli Nord.

però, si sono spostati poco lontano, praticamente dietro casa mia. Quindi, posso testimoniare con quasi matematica certezza che il problema è stato solo spostato. Oltre al problema dei rom, c'è questo continuo sversamento di rifiuti su tutte le strade, anche sull'Asse mediano, sempre in quelle zone, dove, praticamente, non c'è la possibilità di intervenire, se non aspettando che qualcuno passi passi e, nel giro di pochi secondi, inneschi un incendio. Poi, nel momento in cui arrivano i Vigili, è troppo tardi. L'unica nota positiva è che, quando viene a piovere,

quando a me risulta che non vengono monitorati inquinanti come diossine e furani, che sono quasi sicuramente presenti nel *fallout* di ricaduta degli incendi. Non capiamo, dunque, perché l'ARPA non faccia questo tipo di analisi,

Signor Presidente, con riferimento all'atto parlamentare della senatrice De Petris, inerente i comportamenti discriminatori posti in essere da un datore di lavoro nei confronti di un lavoratore affetto da grave disabilità, passo ad illustrare quanto segue. L'articolo 3 della Costituzione enuncia il principio di uguaglianza, riconoscendo a tutti i cittadini pari dignità sociale e uguaglianza: «davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Tale principio si riferisce a tutti i cittadini in quanto tali e non già in relazione all'attività lavorativa svolta. Il comma 2 dell'articolo 15 della Statuto dei lavoratori, come modificato dal decreto legislativo n. 216 del 2003, prevede invece una specifica forma di tutela contro gli atti e i patti discriminatori, ivi inclusi quelli per motivi di *handicap*, posti in essere dai datori nei confronti dei lavoratori. Tra gli altri provvedimenti legislativi in materia di garanzia contro le discriminazioni, vanno ricordati i decreti legislativi nn. 215 e 216 del 2003, con i quali vengono tutelate, rispettivamente, la parità di trattamento fra persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Tali decreti hanno una struttura comune, ma diverso campo di applicazione: il decreto n. 216 riguarda, infatti, specificamente l'accesso al lavoro e l'occupazione. n. 216 del 2003, in particolare, tutela tra l'altro l'accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente; l'occupazione e le condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni di licenziamento; l'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali. L'articolo 2 fornisce la nozione di discriminazione, distinguendo tra diretta e indiretta, mentre per quanto riguarda l'ambito soggettivo, il decreto n. 216 del 2003 tutela il lavoratore, sia esso subordinato, autonomo o parasubordinato. Per quanto concerne la tutela giurisdizionale dalle discriminazioni in parola, il decreto legislativo n. 216 del 2003 rinvia al rito disciplinato dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011 mediante il quale è possibile rivolgersi al tribunale per ottenere la cessazione del comportamento del comportamento pregiudizievole e l'adozione di un comportamento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione accertata, oltre che, se del caso, il risarcimento del danno. Preciso inoltre che la legittimazione ad agire è attribuita al lavoratore che ha subito la discriminazione, nonché alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni ed organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso. Ricordo altresì che la legge n. 67 del 2006, recante misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità. Tale legge precisa che nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro valgono le disposizioni del citato decreto legislativo n. Per quanto concerne le iniziative che il Ministero del lavoro può intraprendere in tale ambito, preciso che le direzioni territoriali del citato Ministero possono effettuare, su richiesta del lavoratore che lamenta una discriminazione a causa del sua disabilità, accertamenti tesi ad acquisire elementi probatori utilizzabili dal medesimo lavoratore nelle competenti sedi giudiziarie. Infine, per quanto concerne il caso del lavoratore menzionato nell'atto parlamentare in parola, la direzione territoriale del lavoro di Roma ha reso noto che la vicenda è stata definita con verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti presso il tribunale di Roma l'11 giugno 2015.

Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per l'elenco di tutti i sistemi e delle norme che presiedono

è accaduto moltissime altre volte, vi era stato un pronunciamento del giudice del lavoro, che aveva, tra l'altro, dichiarato il provvedimento

a tutela dei diritti dei lavoratori e antidiscriminatorio - si è, a nostro avviso, fortemente indebolito (anche a causa del clima politico che si respira),

Signor Presidente, passo ad illustrare l'atto parlamentare del senatore Barozzino concernente il Centro oli e gas "Tempa Rossa" di Corleto di Perticara. Al riguardo, fornisco gli elementi informativi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria compiuta dal Ministero che rappresento. Innanzitutto premetto che le attività di accertamento ispettivo da parte della competente direzione territoriale del lavoro non sono ancora concluse a causa della complessità del cantiere, caratterizzato dalla frammentazione delle attività in opera affidate in subappalto a diverse imprese. Il progetto complessivo relativo alla costruzione del Centro oli e gas "Tempa Rossa", situato nel Comune di Corleto di Perticara, è stato, infatti, affidato dalla società petrolifera Total alla tra la SpA Tecnimont e la SpA KT quali appaltatore e contraente generale per la progettazione, fornitura dei materiali, costruzione ed avviamento dell'impianto, che si servono di una filiera di appaltatori per le diverse strutture. Alla data dell'accesso ispettivo della direzione territoriale del lavoro, il 9 agosto scorso, erano presenti 1.852 unità di cui 1.557 italiane e 295 straniere. Rispetto al totale dei 1.852, 407 sono risultati i lavoratori somministrati da agenzie interinali, 54 distaccati da altre imprese, mentre 10 sono i lavoratori autonomi. Inoltre la percentuale dei lavoratori stranieri attualmente è risultata pari al 16 In ogni caso, le cifre riguardanti l'impiego di personale sul cantiere sono verificabili, settimana per settimana, e comunicate alla competente prefettura ai fini antimafia. Faccio presente, inoltre, che il responsabile della società petrolifera Total ha sottolineato l'attenzione della stessa al rispetto delle norme in materia ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro inserite nei contratti sottoscritti con le imprese appaltatrici. La Regione Basilicata, interpellata al riguardo, ha riferito che lo scorso 29 giugno, su richiesta delle organizzazioni sindacali, si è tenuto, presso la presidenza della Regione, un incontro tra organizzazioni sindacali, La Regione Basilicata ha comunicato di aver ricevuto, nel corso della riunione, rassicurazioni sulla volontà di verificare ogni opportunità utile alla continuità lavorativa dei contratti in scadenza o recentemente scaduti, nei limiti del possesso, da parte dei lavoratori interessati, delle mansioni necessarie per le lavorazioni richieste. Inoltre, è stato assicurato alla Regione e alle organizzazioni sindacali un successivo approfondimento ricognitivo, a cura delle stesse imprese presenti al tavolo di discussione, volto alla esatta verifica della consistenza di manodopera straniera al momento impiegata e di lavoratori residenti nelle zone limitrofe al Centro oli o comunque in Basilicata. Segnalo, inoltre, che la Regione Basilicata ha sollecitato l'istituzione di un tavolo di discussione tra le organizzazioni sindacali e le imprese operanti, demandando a quest'ultimo la gestione delle problematiche in parola. Da ultimo, voglio sottolineare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a seguire la vicenda, anche alla luce degli esiti delle verifiche ispettive ancora in corso.

con le stesse mansioni e con l'aggravante che, mentre i lavoratori italiani prendono 9 euro ad ora, i lavoratori stranieri ne prendono 5. Inoltre fanno degli orari totalmente diversi e non hanno nessun contatto con i lavoratori italiani, quindi non si parlano tra di loro.

Speriamo che, con l'ulteriore accertamento che lei ha detto di voler effettuare, questa sia la volta buona per dare delle risposte. Va inoltre accertato (perché anche questo riferiscono le miei fonti) l'aspetto sanitario in cui vivono i lavoratori stranieri,

Ripeto: non parliamo di lavoratori che vanno a svolgere una mansione diversa o più gravosa, ma di lavoratori che sostituiscono altri lavoratori. È quanto di più meschino può succedere nel mondo del lavoro.

la salute*. In merito al quesito posto dall'interrogazione in esame, si rappresenta che il sale alimentare è definito all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 106 del 31 gennaio 1997 (concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare) come il prodotto ottenuto - cito - dall'acqua di mare, dai giacimenti salini sotterranei oppure dalle salamoie naturali. Lo stesso decreto stabilisce che il sale ottenuto come sottoprodotto da procedimenti industriali non può essere destinato all'alimentazione umana. Ai sensi dell'articolo 3 del suddetto regolamento il sale alimentare deve contenere: non meno del 97 per cento di cloruro di sodio calcolato su sostanza secca; non più dello 0,5 per cento di sostanze insolubile in acqua calcolate su sostanza secca; non più dello 0,3 per cento di sostanze insolubile in acido cloridrico (0,1) calcolate su sostanza secca, e non deve contenere contaminanti in quantità tali da costituire pericolo per la salute. Il sale alimentare può contenere alcuni costituenti secondari naturali in quantità variabili in funzione dell'origine e del metodo di produzione (per esempio, solfati, carbonati, bromuri di calcio, di potassio, di magnesio e di sodio, nonché cloruri di calcio, potassio e ancora magnesio). L'articolo 5 del citato regolamento detta anche le disposizioni in materia di etichettatura; questa deve riportare le seguenti indicazioni: (acqua di mare, giacimenti sotterranei, salamoia naturale) e la specificazione relativa alla forma di presentazione (sale fino o sale grosso). Recentemente l'Organizzazione mondiale per la salute ha raccomandato per la popolazione adulta un consumo di cloruro di sodio inferiore a 5 grammi al giorno (equivalenti a 2 grammi al giorno di sodio). Il sale prodotto da generici processi industriali di ricristallizzazione determinerebbe, secondo le informazioni trasmesse, una purezza (percentuale di cloruro di sodio) pari al 99,9 per cento rispetto ad un sale alimentare che presenti una purezza pari ad almeno il 97 per cento (minore tenore su sostanza secca previsto dal decreto); un sale con questo tenore risulterebbe in ogni caso conforme, in termini di titolo di cloruro di sodio, a quanto indicato all'articolo 3 del sopracitato decreto. In ogni caso, è opportuno sottolineare che le diversità delle materie prime impiegate rende i sali alimentari disponibili inevitabilmente caratterizzati da naturali oscillazioni in termini di tenore di cloruro di sodio. l'incremento ipotetico di esposizione al sodio attraverso il consumo di un sale alimentare caratterizzato da un contenuto superiore al limite minimo previsto dalla legge (in ogni caso un contributo aggiuntivo massimo pari al 3 per cento) non sembra essere significativo. Si sottolinea, inoltre, che il gusto del sale naturale è correlabile alla sua composizione che, per natura stessa del prodotto, può differire sia in termini qualitativi (per profilo compositivo) sia in termini di concentrazione. Non sembra, pertanto, possibile correlare automaticamente e oggettivamente il gusto di un sale alimentare con la sua composizione naturale, peraltro caratterizzata da variabilità dipendente dalla tipologia di produzione. Infine, per quanto riguarda la problematica inerente al sale ricristallizzato, si sottolinea che il sale, per essere destinato ad uso alimentare, deve comunque e sempre rispettare quanto previsto

Mentre infatti la prima parte della risposta dà atto della normativa, che peraltro è stata abbondantemente citata nell'interrogazione, si tralascia sostanzialmente di rispondere sul tema

La questione fondamentale, a nostro avviso, è che la normativa vigente non prevede una corretta, completa e compiuta informazione al cittadino utente, al consumatore. Il consumatore ha diritto di sapere quando compra una confezione esattamente che cosa sta comprando, da dove origina il prodotto e come il prodotto è stato ottenuto e lavorato.

rappresenta una componente fondamentale per il buon funzionamento della rete trapiantologica nazionale e della gestione dell'evento «donazione trapianti»,

la perdita di organi registrata è stata causata essenzialmente da una non corretta conservazione degli organi o per trasporti effettuati con tempistiche non adeguate ai tempi per mantenere l'idoneità dell'organo al trapianto. In particolare, l'accordo mira a fornire indicazioni relative a *standard* operativi per il trasporto in sicurezza sia degli organi, sia delle *équipe* trapiantologiche, sia dei materiali biologici per la conservazione, il ricondizionamento ed il trasferimento di organi per il trapianto, al fine di assicurare un livello di qualità uniforme e rilevabile su tutto il territorio nazionale, nonché un sistema di controllo ed il contenimento dei costi in questa attività. A tal fine, per assicurare un'uniformità sul territorio nazionale e, quindi, l'armonizzazione dei modelli di trasporto attualmente adottati a livello regionale, si è individuata la rete del sistema di emergenza territoriale «118» come riferimento organizzativo.

dell'organo durante il trasporto, prevedendo la definizione, con accordo Stato-Regioni, di specifiche procedure operative volte a garantire l'integrità dell'organo durante il trasporto. In particolare, con l'accordo sono state fornite alle Regioni e alle Province autonome le indicazioni organizzative che consentono di uniformare il modello di trasporto adottato e sono stati fissati i requisiti tecnici e le procedure operative per confezionamento, contenitori, etichettatura, monitoraggio della temperatura e tracciabilità di posizione e temperatura dell'organo, atti a garantire la conservazione e la tracciabilità dell'organo (che deve essere univocamente identificato e riconoscibile a partire dalla sala di prelievo e sino alla sala di trapianto, in ogni fase del trasferimento, inclusi i periodi di immobilità), e assicurare il controllo dei tempi e la sicurezza del trasporto. Inoltre, al Centro nazionale trapianti è affidata la sorveglianza sulla rete nazionale dei trasporti e di coordinamento operativo della stessa attività. stante le stringenti misure adottate con l'accordo, con le quali si sono elevati gli *standard* di qualità e sicurezza del trasporto degli organi, e considerato che l'evento donazione-trapianto non è programmabile

Conosco molto bene l'accordo della Conferenza Stato-Regioni che, tra l'altro, ci ha collocato nel panorama europeo tra i primi Paesi e, come punto di riferimento per il tipo di accordo prestato, per i requisiti posti in essere e per la consapevolezza della nostra capacità di rete e di protezione dell'organo.

Lei, alla fine della sua risposta, ha sottolineato il fatto che proprio per l'imprevedibilità dell'espianto di un organo per un terrorista sarebbe difficile pianificare. Nelle pieghe dell'impossibile si annida anche il possibile, tant'è che uno di questi involucri non tracciati è stato utilizzato, attraverso un'ambulanza, per il trasporto di stupefacenti.

rimane sempre una piccola sacca di Regioni che non si stanno adeguando a delle norme che, tra l'altro, sono state sancite e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni. conclusione, la ringrazio per la risposta, che è stata assolutamente pertinente e completa, però le chiedo di verificare e controllare le Regioni che non si attengono a una normativa che ormai ha più di un anno di vita.

Signor Presidente, l'interrogazione della senatrice De Petris, concerne l'operazione di dismissione in favore del Fondo immobili pubblici, la gestione degli immobili dismessi e le relative modalità di vendita poste in essere dal citato fondo. L'operazione di dismissione, avviata nel 2004, ha interessato un portafoglio di 396 immobili, appartenenti per il 70 per cento alle amministrazioni centrali e per il restante 30 per cento agli enti previdenziali INPS, INAIL e INPDAP ed è stata strutturata finanziariamente in due distinte *tranche*: la prima, di ammontare pari al 40 per cento del totale, finanziata tramite l'emissione di quote; la seconda, pari al restante 60 per cento del valore complessivo degli immobili, realizzata tramite un finanziamento contratto dal Fondo con un gruppo di banche riunite in consorzio. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 9 giugno 2004 (cosiddetto decreto di avvio dell'operazione), il Ministero dell'economia e delle finanze ha selezionato con procedura competitiva le banche e gli istituti finanziari di comprovata esperienza nella costituzione del suddetto Fondo immobiliare e nel collocamento delle quote emesse dallo stesso. Tali banche ed istituti hanno assistito il Ministero dell'economia e delle finanze nelle attività relative alla costituzione del Fondo, curando, tra l'altro, la selezione, con procedura di evidenza pubblica, di Investire Immobiliare, quale SGR avente la gestione del Fondo. Detti immobili sono stati ceduti (tramite decreto di apporto 23 dicembre 2004 e due decreti interministeriali di trasferimento di pari data, tutti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2004, n. 303)

Nell'ambito dell'operazione descritta, all'Agenzia del demanio è stato affidato il ruolo di conduttore unico. I rapporti intercorrenti tra il Fondo immobiliare e l'Agenzia (oltre che tra la stessa Agenzia e le amministrazioni assegnatane) sono stati regolamentati sulla base delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 15 dicembre 2005, (Fondo immobili pubblici: decreto operazione) e successivamente recepite dal contratto di locazione stipulato dall'Agenzia del demanio con il Fondo e dai

non incide su obiettivi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico poiché si tratta di immobili ormai di proprietà di privati. Nell'interrogazione viene tra l'altro criticata la scelta del Fondo di una vendita cielo-terra in luogo di una vendita frazionata dei vari complessi immobiliari, laddove il frazionamento avrebbe invece favorito l'esercizio del diritto di opzione e/o prelazione da parte dei conduttori delle unità in locazione passiva. L'immobile in questione, sito in Roma, Piazza Augusto Imperatore, rientra tra quelli oggetto dell'operazione di dismissione immobiliare a favore del Fondo immobili pubblici, ai sensi del decreto-legge del 25 settembre 2001, n. 351. Il Fondo immobiliare chiuso (FIP) è stato costituito in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge del 25 settembre 2001, n. 351, nel quadro di un'operazione di dismissione di immobili pubblici (ad uso diverso da quello residenziale) strutturata secondo lo schema del cosiddetto *sale and lease back*. Ai sensi del successivo decreto ministeriale del 9 giugno 2004 (il cosiddetto e già ricordato "decreto di avvio" dell'operazione), il Ministero dell'economia e delle finanze ha selezionato con procedura competitiva le banche e gli istituti finanziari di comprovata esperienza nella costituzione del suddetto Fondo immobiliare e nel collocamento delle quote emesse dallo stesso. Tali banche ed istituti hanno assistito il Ministero dell'economia e delle finanze nelle attività relative alla costituzione del fondo, curando, tra l'altro, la selezione, con procedura di evidenza pubblica, di "Investire immobiliare". Detti immobili, di proprietà dello Stato e di alcuni enti pubblici (INPS, INPDAP, INAIL), sono stati ceduti alle amministrazioni che li avevano precedentemente in uso. Pertanto l'Agenzia del demanio è conduttrice unica di tutti gli immobili del compendio FIP, mentre le amministrazioni utilizzatrici sottoscrivono con detta Agenzia i disciplinari di assegnazione, i quali riproducono gli obblighi gravanti sull'Agenzia in virtù del contratto di locazione sottoscritto dalla stessa. Ai sensi dell'articolo 17 del contratto di locazione, è previsto, nei casi di vendite di singoli immobili da parte di FIP, il diritto di prima offerta a favore dell'Agenzia del demanio che, per sé o per conto delle amministrazioni utilizzatrici interessate, potrà riacquistare l'immobile con prelazione rispetto a possibili terzi acquirenti. Inoltre, per quanto riguarda la pretesa titolarità di un diritto di prelazione e/o opzione, ai sensi dell'articolo 3 del più volte richiamato decreto-legge n. 351 del 2001, si evidenzia che tale pretesa non può trovare fondamento nel caso di specie, in quanto: innanzitutto, tutti gli immobili del compendio FIP, compresi quelli gravati da vincolo di interesse culturale (tra cui l'immobile di Roma, Piazza Augusto Imperatore, oggetto di uno dei quesiti dell'interrogazione), rientranti nel decreto interministeriale 23 dicembre 2004, furono apportati o trasferiti attraverso una cosiddetta vendita in blocco, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legislativo inoltre, la previsione del diritto di opzione-prelazione in favore del conduttore, di cui all'articolo 3 (e non 4), fa riferimento ai casi di privatizzazione mediante cessione di immobili a società veicolo. Il caso in esame, invece, come abbiamo sottolineato, riguarda la dismissione di immobili a fondi comuni di investimento immobiliare, disciplinata ai sensi dell'articolo 4. Le due forme dì privatizzazione sono in realtà ben diverse: la cessione di immobili a società veicolo (*ex* articolo 3) integra un'ipotesi di vendita cumulativa in cui viene fatto salvo il diritto di opzione e successiva prelazione in favore dei conduttori (residenziali e non). Nel passato, per tale tipologia di dismissioni sono stati emanati decreti ministeriali che nel dettaglio hanno disciplinato le modalità di esercizio dell'opzione e prelazione a favore dei conduttori. Nella dismissione a favore di un fondo immobiliare costituito dallo Stato (*ex* articolo 4), l'operazione è invece più complessa e la vendita e strutturata come cosiddetta vendita in blocco. Pertanto, conformemente agli orientamenti giurisprudenziali su tali tipologie di vendite, non è esercitabile per alcun tipo di immobile un diritto di opzione-prelazione in favore dei pregressi conduttori. Ciò perché: in primo luogo, il conduttore unico dell'intero compendio è, *ex lege*, l'Agenzia del demanio; luogo, solamente l'Agenzia, allorquando il singolo fabbricato sarà messo in vendita dal fondo (e perciò potrà allo stesso essere riconosciuta un'autonomia diversa dall'intero compendio trasferito), potrà esercitare il diritto di prelazione direttamente o indirettamente (per se stessa o per conto di altra amministrazione utilizzatrice dell'immobile messo in vendita), così come previsto nel cosiddetto decreto operazione, precedentemente richiamato, e nel contratto di locazione tra l'Agenzia del demanio e FIP. Nel caso dell'immobile di Roma, sito in Piazza Augusto Imperatore, i conduttori citati nell'interrogazione (il ristorante "Gusto" e il negozio "Dentice"), non avevano pertanto un diritto di opzione-prelazione legale al momento della vendita dell'immobile a favore del fondo, e non ce l'hanno oggi che il fondo ha messo in vendita l'immobile, essendo subconduttori rispetto al contratto stipulato con l'Agenzia del demanio. Si fa presente inoltre, che, diversamente da quanto asserito dall'interrogante, le operazioni di vendita poste in essere dai Fondi immobili pubblici non prevedono alcun tipo di valutazione concertata preventivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine all'effettiva opportunità o modalità di vendita di un determinato immobile, essendo il Fondo un soggetto privato che agirà nell'interesse dei quotisti. Inoltre, gli immobili, una volta conferiti-trasferiti ai Fondi, diventano proprietà privata degli stessi e di conseguenza le vendite non incidono, come ricordato, sul raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio immobiliare o sugli equilibri di finanza pubblica. E ancora, uno dei compiti istituzionali della direzione VIII del dipartimento del tesoro è la gestione delle attività connesse e strumentali a operazioni di valorizzazione e dismissione di beni immobili, nell'ambito dei fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 410 del 2001, ma in dette attività non rientra in alcun modo il monitoraggio sulle tempistiche delle dismissioni operate dai Fondi immobiliari in favore dei terzi acquirenti se non per gli impegni contrattualmente assunti a carico dell'Agenzia del demanio ovvero a carico del Ministero stesso. Infine, per quanto riguarda le attività volte a minimizzare gli impatti negativi della ricordata operazione avviata nel 2004, si aggiunge che, nell'ambito dell'attività dell'Agenzia del demanio, vi è la facoltà di recedere dal contratto di locazione per singoli immobili, riducendo così la spesa complessiva di fitto passivo del compendio conferito ai Fondi. Tale recesso è tuttavia contrattualmente limitato a un numero di immobili i cui canoni siano pari complessivamente al 20 per cento del canone dell'intero compendio per quanto riguarda il FIP, e al 10 cento per quanto riguarda il Fondo Patrimonio 1. L'Agenzia, in base alla pianificazione finora effettuata, volta a una gestione attiva di minimizzazione degli impatti negativi sul conto economico dello Stato, ha sostanzialmente esaurito le citate percentuali di recesso disponibili,

sono già in via di esercizio i recessi per il ridotto numero di immobili, già peraltro individuati, ai quali era applicabile la residua (ormai molto bassa) percentuale di recesso:

si evidenzia altresì che l'Agenzia, in vista della scadenza dei contratti di locazione con i Fondi (dicembre 2022 per il FIP e dicembre 2023 per il Fondo patrimonio 1) sta predisponendo, di concerto con tutte le pubbliche amministrazioni utilizzatrici degli immobili e su indicazione del dipartimento del Tesoro, un piano d'azione finalizzato al rilascio di tutti gli immobili entro un anno dalle citate scadenze contrattuali, sempre al fine di ridurre la spesa pubblica per fitto passivo. La definizione di tale piano è tuttavia caratterizzata dalla necessità di individuare soluzioni allocative alternative per tutti gli uffici utilizzatori tra cui quelli con particolari esigenze ubicazionali, dimensionali e impiantistiche, tali da rendere "strategici" gli immobili di proprietà dei Fondi attualmente in uso, e pertanto potenzialmente non rilasciabili. Il numero provvisorio di tali immobili "strategici", variabile in funzione delle interlocuzioni in corso con le varie pubbliche amministrazioni utilizzatrici, è ad oggi pari a 113 immobili su un totale di 341 condotti in locazione al 1° semestre 2016.

che nella legge fosse molto ben chiaro il diritto di opzione. Tale diritto, all'inizio proprio in quest'Aula del Senato, fu introdotto, non soltanto per i conduttori privati, in caso di vendita in blocco, ma anche per gli esercizi commerciali.

degli introiti e delle risorse, perché è un fatto incredibile: è come se io possiedo una casa, ci abito, a un certo punto decido di venderla, la do a

per contribuire al risanamento della finanza pubblica, forse è arrivato il momento di fare un bilancio e considerare ciò che effettivamente è entrato e quali sono stati i vantaggi. Nello specifico,

rientrano nell'ambito dell'operazione "bastabuchesullestrade", con la quale la società ha avviato un vasto progetto di manutenzione straordinaria della rete stradale di competenza sull'intero territorio nazionale. In particolare, per la strada statale n. 1 Aurelia sono stati previsti, in una prima *tranche*, sette interventi di risanamento profondo della pavimentazione, con stabilizzazione della fondazione stradale della corsia di marcia e successiva ricostruzione del pacchetto bituminoso per l'intera carreggiata, con stesa di tappeto drenante. Nell'ambito dei lavori avviati con le risorse messe a disposizione nel contratto di programma 2015, sono stati completati i seguenti interventi: il primo, avviato lo scorso giugno, ha riguardato la tratta compresa dal chilometro 238 al chilometro 240 in carreggiata nord nel Comune di Piombino, tra gli svincoli di Riotorto e Venturina, con apertura al traffico in data 2 luglio 2016; il secondo, avviato sempre nello scorso mese di giugno, è stato effettuato dal chilometro 208 al chilometro 210, in carreggiata sud nel Comune di Grosseto, tra gli svincoli di Gavorrano e Giuncarico, con apertura al traffico il successivo 15 luglio scorso; il terzo, dal chilometro 265 al chilometro 268 in carreggiata Nord nel Comune di Castagneto Carducci, tra gli svincoli di Donoratico e Cecina Sud, è stato avviato l'11 luglio 2016 e l'andamento dei lavori di risanamento della pavimentazione stradale ha consentito la completa rimozione del cantiere il successivo 21 luglio. Nel suddetto tratto, infatti, completati i prioritari interventi idonei a garantire le necessarie condizioni di sicurezza e percorribilità dell'arteria, è stata ripristinata la circolazione su entrambe le corsie disponibili per le due direttrici di marcia, mantenendo, solo sulla carreggiata nord, dal chilometro 266 al chilometro 268, la limitazione di velocità di 50 chilometri Gli interventi di completamento concernenti la stesa del tappeto drenante sono stati posticipati al fine di agevolare i flussi di traffico del periodo estivo, in accordo con quanto auspicato dall'assessorato alle infrastrutture della Regione Toscana e richiesto dai Comuni di Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci e San Vincenzo; il completamento è previsto per il prossimo 23 settembre. ANAS ha inoltre fornito le seguenti notizie sui restanti quattro interventi. Il quarto intervento ha interessato il tratto compreso tra il chilometro 315+790 e il chilometro 318+100, in carreggiata nord nel Comune di Livorno. I lavori, tra il tratto dal chilometro 315+790 e il chilometro 317+319, iniziati il 18 luglio scorso, sono stati sospesi il successivo 21 luglio con riapertura al traffico su entrambe le carreggiate; tali lavorazioni sono state, quindi, riprese lo scorso 5 settembre e ultimate il 9, data dalla quale il tratto è stato riaperto al transito. Dal prossimo 28 settembre al 6 ottobre 2016, è prevista l'estensione del suddetto intervento sino al chilometro 318+950, con la sola parzializzazione della carreggiata. Il quinto riguarda il tratto compreso tra il chilometro 217+900 e il chilometro 219+500 in carreggiata nord nel Comune di Scarlino, tra gli svincoli di Gavorrano e Scarlino; i lavori hanno avuto inizio il 5 settembre, con ultimazione prevista entro il corrente mese. Il sesto riguarderà il tratto compreso tra il chilometro 281 e il chilometro 283+590, in carreggiata nord nel Comune di Cecina, tra lo svincolo di Cecina Centro e la barriera del Casello di Rosignano dell'Autostrada SAT; i lavori avranno inizio il prossimo 1° ottobre, con ultimazione prevista per il 21 dello stesso mese. Il settimo e ultimo intervento riguarderà il tratto compreso tra il chilometro 259+900 e il chilometro 261, in carreggiata nord nel Comune di San Vincenzo, tra gli svincoli di Donoratico e Cecina Sud; i lavori avranno inizio il 24 ottobre prossimo con ultimazione prevista il successivo giorno 28. È stato altresì attivato un ulteriore intervento che riguarderà il rifacimento della pavimentazione nel tratto compreso tra il chilometro 188+300 e il chilometro 191+400, in carreggiata nord nel Comune di Grosseto,

dal mese di ottobre sono programmati interventi di ripristino della pavimentazione ammalorata sulle rampe degli svincoli di Cecina Nord, Cecina Centro, Cecina Sud-la California e Donoratico nel Comune di Castagneto Carducci

In primo luogo, perché è stato quantomeno anomalo aver presentato un atto ispettivo in ragione dell'avvio di cantieri di lavoro, quando normalmente è prassi inveterata che è la mancanza del loro avvio a costituirne il presupposto. In secondo luogo, luogo, capisco che è stato singolare avere comunque voluto mantenere l'atto ispettivo, ovvero l'interrogazione, nonostante questa avesse già sortito il suo effetto, inducendo il il cambiamento in un atteggiamento da parte del direttore dei lavori che aveva finito per costituire - questo sì - il vero problema della situazione che si era determinata. Tutto ciò mi consente di di ringraziarla, oltre che per la tempestiva attivazione della struttura ministeriale e dell'ANAS, anche per la prontezza con cui è venuto a darne conto in Parlamento. Parlamento. Tuttavia, nonostante l'apprezzamento anche per il dettagliato lavoro che ci ha rappresentato in corso dal punto di vista degli interventi manutentivi di ANAS, ritengo che il tema sollevato non sia stato assolutamente peregrino e che mantenga

casi analoghi - riguarda l'avvio di lavori di manutenzione straordinaria significativi e importanti come quelli sulle strade statali statali - nel caso specifico, l'Aurelia - che, con il loro attraversamento di alcuni Comuni (nel caso della Provincia di Livorno, Comuni costieri), di fatto ne costituiscono l'unica arteria di scorrimento. La forte e, per certi versi, inevitabile limitazione della viabilità per i lavori programmati rischiava, nel caso specifico, di compromettere l'attività di molti operatori economici e lavoratori stagionali; più in generale, ovviamente, essa dà luogo a disagi non sempre giustificati e giustificabili alla popolazione, soprattutto in un momento di particolare intensità turistica, come nel caso da lei indicato.

un intervento che ragionevolmente non aveva i presupposti dell'emergenza e dell'urgenza e per il quale si accampava una ragione di stagionalità. Mi fermo qui. Credo che

e di sollecitare un'attenzione maggiore rispetto alle sensibilità e alle esigenze economiche di un territorio e di una comunità che, in un momento come quello attuale, in cui persiste una seria crisi economica, sono sicuramente interessati alla realizzazione dell'intervento, ma non certo a pagarne un prezzo sicuramente eccessivo. La ringrazio comunque per la più che esauriente risposta e per l'aggiornamento sullo stato dei lavori in corso.

in relazione ai quesiti posti, gli uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiariscono, preliminarmente, che le verifiche periodiche e l'eventuale taratura dei dispositivi per l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità sono già previste, con un regime diverso secondo se utilizzati in modalità automatica non presidiata o sotto il diretto controllo degli organi di polizia. Nel primo caso, già dal 2004, anno delle prime approvazioni di dispositivi totalmente automatici da utilizzare senza il presidio della polizia, le verifiche periodiche sono state previste con cadenza almeno annuale, così come riportato dai decreti di approvazione e nei manuali d'uso; mentre per i dispositivi gestiti direttamente dagli operatori di polizia i controlli da eseguire sono previsti nei manuali d'uso e manutenzione. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015, si rende necessario modificare l'articolo 45, comma 6, del vigente codice della strada, nel senso indicato dalla Corte medesima. Ed infatti, i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, proprio al fine dell'adeguamento alla citata sentenza, stanno svolgendo un'attività di ricerca e di approfondimento per prevedere l'obbligo, attraverso apposito decreto ministeriale, di controlli e verifiche periodiche per i dispositivi direttamente gestititi dagli organi di polizia stradale, come per quelli totalmente automatici, così da uniformare le procedure. Circa il corretto utilizzo dei dispositivi rilevatori di velocità, il Ministero dell'interno, che coordina i servizi di polizia stradale da chiunque svolti a norma dell'articolo 11 del codice della strada, riferisce di prestare da tempo notevole attenzione alla tematica della piena e continuativa funzionalità di tali apparecchiature, già in epoche precedenti la citata sentenza n. 113 della Consulta. Infatti, la competente direzione centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza ha fornito specifiche direttive in materia alle articolazioni territoriali del servizio di polizia stradale. In particolare, con la circolare del 13 dicembre 2013, emanata congiuntamente con la direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in mancanza di un generalizzato obbligo di taratura, si è ribadita la necessità, per gli organi di polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento e l'osservanza dei limiti di velocità, di rispettare le modalità di installazione e di impiego previste dai manuali d'uso e, quindi, anche l'obbligo della verifica periodica dell'apparecchiatura in esame. Il Ministero dell'interno precisa altresì che la verifica, di norma, è prescritta nel decreto di approvazione del singolo apparecchio, qualora questo sia destinato ad essere utilizzato in modo completamente automatico, cioè senza la presenza di un operatore di polizia stradale. Per quanto concerne, invece, le apparecchiature destinate ad essere impiegate esclusivamente con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia stradale, con circolare del 26 giugno 2015 direzione centrale, allo scopo di consentire il rispetto dei principi enunciati dalla Corte costituzionale, ha invitato le articolazioni territoriali a non utilizzare le citate apparecchiature, se non prima di averle sottoposte a verifica periodica di funzionalità. Al riguardo, corre l'obbligo di precisare che in genere i decreti di approvazione non prevedono una verifica periodica di funzionalità per quest'ultima tipologia di apparecchiature. Ciò in quanto le stesse sono dotate di sistemi di autodiagnosi dei guasti e la relativa funzionalità è verificabile dall'operatore stesso prima di iniziare l'attività di controllo; si tratta in particolare dei dispositivi denominati Telelaser (in tutte le versioni) e Provida. Per quanto riguarda specificamente la Provincia di Padova, il compartimento della polizia stradale per il Veneto ha riferito che, dopo la citata sentenza, tutte le apparecchiature in uso presso le proprie strutture territoriali per il rilevamento delle violazioni ai limiti di velocità sono state fermate e inviate presso un centro accreditato dal Sistema nazionale di taratura. Quanto agli otto autovelox in dotazione al Comune di Padova, l'amministrazione locale ha comunicato che per gli stessi è prevista da contratto una manutenzione ordinaria annuale di taratura, di certificazione del sistema e di monitoraggio tecnico.

Ma, vede, la sicurezza delle persone nella circolazione stradale rientra tra le finalità primarie perseguite dallo Stato: lo dice l'articolo 1, comma 1, del codice della strada. Cioè la legge prescrive, anche nel testo seguente e nelle normative seguenti, che gli autovelox fissi debbano essere installati per garantire la sicurezza su strade critiche e con particolare frequenza di incidenti e dove sia documentata l'impossibilità o la difficoltà di procedere alla contestazione immediata. Servono dunque uno studio che includa la localizzazione esatta del tratto, la sua descrizione accurata (con documentazione fotografica, disegni, piantine e planimetrie), i dati sul traffico (quali e quanti veicoli transitano), sul numero di sinistri negli ultimi cinque anni (con quali conseguenze e quali cause presumibili) eventuali difficoltà operative nel procedere alla contestazione immediata. Poi serve il parere dell'ente proprietario della strada circa la compatibilità tecnica dell'installazione con la fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione. Il prefetto, a questo punto, valuta l'esistenza della congruità degli atti e identifica dove effettivamente è possibile installare autovelox. Servono poi una serie di altre condizioni. Vanno rispettate, a tutela del cittadino, le garanzie sulla corretta omologazione, l'autorizzazione, l'installazione secondo norma e le regolari tarature e manutenzioni. Aggiungiamo che gli autovelox devono essere anche visibili e correttamente segnalati, altrimenti non servono a fare sicurezza. Il cittadino che vede un dispositivo all'ultimo momento sicuramente avrà una multa, ma non si avrà alcun effetto preventivo sulla sicurezza, anzi, si possono indurre frenate brusche con le conseguenze del caso. Se non ci sono tutte queste condizioni non sono giustificati gli autovelox e si conferma il dubbio che la loro installazione non sia finalizzata alla sicurezza. la questione centrale che le voglio sottoporre è la seguente: chi controlla la correttezza di tutti questi passaggi? Vediamo riportata dalla stampa una enormità di ricorsi.

perché lo Stato ha tagliato i fondi agli enti locali e il cittadino ha l'impressione chiara che in cambio abbia fornito un mezzo per fare cassa determinando un *far west* di abusi. Lo deduciamo dalla stessa legge quando prescrive che la metà delle sanzioni debba essere investita per migliorare la sicurezza - sottolineo: la metà - ammodernando la segnaletica, installando *guard rail* più sicuri e quant'altro ma il resto va a fare cassa e sembra proprio questo l'obiettivo principale. Quanti danni e quanti morti e feriti dobbiamo imputare al fatto che si persegue lo scopo di prelevare denaro in maniera surrettizia, sacrificando il tema della sicurezza? Ci sono poi altre questioni: quanto intasiamo i nostri tribunali a causa di questo *far west*? Ci rimettono le imprese, che vedono nella lentezza del sistema giudiziario un freno allo sviluppo. E poi fare ricorsi costa. Per un cittadino che va fino in fondo e se lo può permettere, ce ne sono altri che rinunciano e pagano. Dovrebbe essere, a nostro avviso, lo Stato, il suo Dicastero a garantire la regolarità di questo sistema e invece la giustizia e la certezza del diritto se la devono pagare privatamente i cittadini. Solo grazie alle loro azioni abbiamo scoperto quali e quanti strumenti erano illegittimi e inefficaci. Allora, per tutte le segnalazioni che riceviamo, signor Sottosegretario, per l'appello di tante organizzazioni di tutela dei cittadini, le ho chiesto, come parlamentare del Movimento 5 Stelle, un tavolo tecnico. L'ho chiesto con urgenza, perché abbiamo una quantità di verifiche da chiedere, ben oltre quelle sulle quali ci ha dato parziali rassicurazioni, e anche una quantità di soluzioni da proporre. Non abbiamo avuto risposta. Ripeto: non abbiamo avuto risposta. Allora rinnovo l'invito, qui, davanti ai cittadini che ci vedono da casa, e le ricordo che laddove la sicurezza viene posta

preliminarmente devo premettere che la gestione delle autostrade Al8 (Messina-Catania e Siracusa-Gela) e A20 (Messina-Palermo) è affidata in concessione al Consorzio per le autostrade siciliane ai sensi della convenzione stipulata il 27 novembre 2000 con ANAS SpA. Successivamente, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 216 del 2011, relativa legge di conversione, e dell'articolo 36, comma 4, del decreto-legge n 98 del 2011, e relativa legge di conversione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è subentrato ad ANAS nelle funzioni di concedente per tutte le tutte le convenzioni di concessione, costruzione e gestione delle autostrade in essere alla predetta data, tra cui anche la suddetta convenzione con il CAS. In merito alle iniziative per verificare In merito alle iniziative per verificare la presenza di gravi inadempienze da parte del concessionario CAS, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è a conoscenza delle criticità esposte dall'interrogante e, com'è noto, già dal 2006 ha avviato una procedura di contestazione nei confronti del CAS per gravi inadempienze alla convenzione. Tale procedura si è conclusa con il decreto interministeriale n. 457 del 5 luglio 2010, che ha disposto la decadenza della concessione assentita al CAS. Tuttavia, tale provvedimento è stato dichiarato nullo con sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa nel 2011. Nel frattempo, i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno proseguito nella propria attività di verifica e controllo dell'operato del Consorzio prevista dalla convenzione, continuando a contestare allo stesso le molteplici «non conformità» periodicamente rilevate sulle autostrade gestite, tramite l'attività di sopralluogo da parte dell'ufficio territoriale competente. In relazione a ciò è stata difatti avviata, nel gennaio 2013, un'ulteriore procedura di contestazione formale per mancati adempimenti contestati, sia di natura tecnica che amministrativa, relativi al quinquennio 2009-2013. La procedura di contestazione è stata successivamente formalizzata in data 4 dicembre 2014 con atto di diffida e messa in mora per un nuovo pronunciamento di decadenza della concessione. A seguito delle controdeduzioni addotte dal Consorzio, le stesse sono state rigettate e, ad oggi, è in fase conclusiva la relativa istruttoria, che potrà produrre una nuova disposizione di decadenza. In aggiunta a tale contestazione formale e per fatti successivi all'avvio della stessa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini del riconoscimento dell'adeguamento tariffario, ha ulteriormente avanzato al CAS contestazioni per inadempimenti di natura tecnica e amministrativa, al 30 giugno dell'anno 2014 (relativi all'anno 2013), al 30 giugno dell'anno 2015 (relativi all'anno 2014) e, da ultimo, al 30 giugno 2016 (relativi all'anno 2015), fornendo quale termine per le controdeduzioni venti giorni, entro i quali il Consorzio non ha risposto, per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procederà ai provvedimenti del caso. Per quanto sopra, in occasione dell'adeguamento annuale delle tariffe autostradali, la cui istruttoria è condotta dalla direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali, al CAS non è stato riconosciuto alcun incremento tariffario a partire dall'anno 2007, proprio per i suddetti inadempimenti amministrativi e contabili. Faccio presente, infine, che il CAS ha aderito all'iniziativa e applica gli sconti per i pendolari regolati dal protocollo di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in base al quale, a partire da febbraio e sino al 31 dicembre 2016, è consentita l'agevolazione tariffaria per i pendolari pari al 20 per cento. Per quanto attiene agli episodi dei sinistri denunciati dall'onorevole interrogante, per l'evento verificatosi nella galleria Battaglia, il competente ufficio di Catania ha espletato all'epoca dei fatti (aprile 2014) le proprie attività di verifica sull'accaduto. Quanto all'incidente verificatosi all'interno della galleria Buonfornello, che insiste su un tratto stradale in gestione ANAS, la stessa società riferisce di aver espletato all'epoca dei fatti le proprie attività di verifica, accertando l'assenza di anomalie connesse all'impianto elettrico presente in galleria ed aggiunge, a puro titolo informativo, che anche l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA Sicilia ha effettuato delle indagini sulla presenza di campi elettromagnetici all'interno del citato tunnel, senza tuttavia rilevare valori anomali rispetto alla media. In merito poi alla mancanza di adeguati sistemi di sicurezza in galleria, evidenzio che anche la Commissione permanente per le gallerie, competente per l'attuazione della direttiva 2044/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete autostradale transeuropea, ha evidenziato la non conformità per quanto riguarda i requisiti minimi di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo n. 264 del 2006, per tutte le 40 gallerie superiori ai 500 metri della rete gestita dal CAS in relazione alle specifiche condizioni riconosciute nel corso delle ispezioni svolte.

Di questo si tratta. Abbiamo contezza dell'assoluta criticità del sistema gestito dal Consorzio per le autostrade siciliane (CAS). In particolare,

che sollecitare il Governo ad eseguire in tempi assolutamente rapidi tutti gli adempimenti necessari per arrivare alla rescissione di tutti i contratti in essere, alla decadenza e a riassumere nella titolarità e nella potestà del Ministero, e conseguentemente, dell'ANAS, di questi importanti tratti autostradali.

Signor Presidente, nel confermare quanto ho premesso nel precedente atto del senatore Mancuso circa la competenza nella gestione delle autostrade A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela e A20 Messina-Palermo, rispondo in merito allo svincolo di Caronia, anche detto di Furiano, posto alla chilometrica 113+500 della A20 Messina-Palermo, che è stato originariamente previsto quale «semi-svincolo provvisorio», a seguito della realizzazione della tratta Sant'Agata di Militello-Furiano. Il semi-svincolo, aperto dal 2002, prevedeva le sole rampe di accesso e di uscita in direzione e provenienza Messina. La barriera fu costruita con elementi e impianti di cui era prevista la riutilizzazione nelle costruende stazioni della successiva tratta Sant'Agata Militello-Cefalù, a dimostrazione del fatto che si trattasse di un'opera che non aveva connotati per costituire un'opera definitiva. L'uscita provvisoria di Caronia fu costruita solo per consentire l'uscita e l'entrata in autostrada da e per Messina. La direttrice per Palermo era in costruzione. Nel marzo 2005 è stata completata e aperta al traffico l'intera tratta Furiano-Castelbuono in entrambe le direzioni e contestualmente è stato reso operativo lo svincolo di Santo Stefano di Camastra, a 21,18 chilometri di distanza dallo svincolo provvisorio di Caronia. Di conseguenza, nel settembre 2007, in concomitanza con l'attivazione degli impianti di esazione della suddetta tratta Furiano-Castelbuono, il semi-svincolo di Caronia è stato definitivamente chiuso dal concessionario CAS e successivamente smontata la barriera provvisoria di esazione del pedaggio. Ad oggi, il semi-svincolo di Caronia, a causa della mancata manutenzione per inutilizzo, presenta condizioni di degrado e una sua riapertura richiederebbe la realizzazione di una nuova stazione di esazione e dei relativi impianti (illuminazione, videosorveglianza nonché un adeguamento alla vigente normativa, considerato anche che la rampa di accesso in direzione Messina si trova in corrispondenza dell'odierna corsia di sorpasso della carreggiata autostradale Palermo-Messina. Infine, secondo il concessionario, il bacino di utenza che potrebbe essere interessato da questa nuova realtà sarebbe quantitativamente limitato e tale da non giustificare la realizzazione dei nuovi impianti.

Intanto devo ricordarle che lo svincolo di Caronia, di cui abbiamo parlato, si trova tra le uscite di Santo Stefano di Camastra e Sant'Agata di Militello, che sono separate da ben 30 chilometri di percorso autostradale.

Bisogna anche considerare che l'uscita di Caronia permette a chi si vuole inoltrare nel Parco dei Nebrodi (uno dei parchi più importanti della Sicilia e credo del'intero Meridione) di accedere più facilmente ad alcuni itinerari e percorsi di quell'area protetta. protetta. Tale svincolo porterebbe quindi a una migliore fruizione di questi luoghi, che sono tra l'altro di rara bellezza e assolutamente suggestivi dal punto di vista naturalistico.

delle potenzialità dello sviluppo turistico di quel territorio. Non mi resta altro che auspicare, nell'ambito di una rivisitazione dei rapporti tra ANAS, Ministero e CAS, facendo anche riferimento alla precedente interrogazione e, quindi, a un'eventuale rescissione di tutti i contratti in essere, ripensamento che possa portare alla riapertura di quello svincolo che, peraltro, già esiste, come lei ha giustamente detto, e che va soltanto riattato.

tengo a precisare che si tratta di interrogazione e interpellanza presentate un anno e mezzo fa e che al momento la situazione è completamente cambiata. Ciò non toglie che la sollecitazione del sottoscritto al Ministero rimane tutt'ora valida, perché l'aumento delle Forze dell'ordine e i maggiori fondi per la videosorveglianza rimangono importantissimi. Le prefetture hanno fatto delle graduatorie per mettere a disposizione i fondi per la videosorveglianza.

marina protetta di Torre Guaceto) è importante che ci siano fondi a disposizione, perché il sistema di videosorveglianza è fondamentale per prevenire furti e rapine.

e che le graduatorie fatte dalla prefettura tempo fa vengano al più presto riviste per mettere a disposizione nuovi fondi.

chiede l'adozione di iniziative volte a sostenere l'azione delle Forze dell'ordine. In particolare, si sollecitano interventi per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza e il potenziamento dei servizi di controllo della compagnia dei carabinieri di San Vito dei Normanni e della stazione dei carabinieri di Carovigno. Va preliminarmente rilevato che tutto il territorio provinciale - non solo quello carovignese - attraversa una fase di effervescenza sotto il profilo sociale, economico e occupazionale con potenziali ripercussioni sull'ordine e sulla sicurezza pubblica, cosa di cui ovviamente il Ministero è consapevole. Nello specifico, il contesto del Comune dì Carovigno si connota per una certa vivacità dei fenomeni di microcriminalità, in particolare di reati contro il patrimonio, in un quadro caratterizzato da una generalizzata negatività delle condizioni economiche e dalla mancanza di concrete occasioni di sviluppo, fattori che concorrono a creare sempre più larghe fasce di disagio sociale ed economico. In tale ambito, si sono registrati anche alcuni episodi di danneggiamento e incendio ai danni di esponenti della precedente amministrazione comunale (rinnovata in occasione delle consultazioni amministrative del maggio 2015), sui quali l'attività infoinvestigativa, coordinata dalla autorità giudiziaria, è stata avviata tempestivamente, sebbene si rilevi a volte una scarsa collaborazione da parte delle vittime. Soggiungo che non si sono registrati casi di dimissioni di amministratori locali eventualmente riconducibili ad atti intimidatori. A seguito degli eventi menzionati, presso la prefettura di Brindisi si sono svolte specifiche riunioni di coordinamento interforze, al fine di acquisire un quadro completo degli elementi utili alla lettura di quanto accaduto. In tali sedi, oltre ad un approfondito esame e monitoraggio di ciascun fenomeno, sono state individuate mirate strategie di prevenzione e repressione, sviluppatesi attraverso una molteplicità di azioni coordinate, per una efficace ed adeguata attività di prevenzione e contrasto rispondente alle esigenze del territorio. L'analisi dell'andamento dei fenomeni delittuosi evidenzia come i reati commessi siano ascrivibili solo in parte alla delinquenza locale. Ed invero in base alle risultanze investigative dell'Arma dei carabinieri è stata rilevata la presenza di criminali provenienti da Comuni limitrofi, i quali, agevolati dall'ottima rete viaria e dalla vastità delle campagne campagne scarsamente popolate e caratterizzate da numerose ville non abitate per la maggior parte dell'anno prediligono il territorio comunale di Carovigno per consumare reati contro il patrimonio. In tale contesto, sebbene i recenti dati statistici relativi al primo semestre di quest'anno, comparati con l'analogo periodo dell'anno scorso, abbiano fatto registrare una significativa flessione dei fenomeni criminosi, permane elevato il livello di attenzione sul territorio di Carovigno, le cui tematiche di rilievo sono state oggetto, anche di recente, di esame nel corso di riunioni di coordinamento interforze. In particolare, il 18 luglio scorso, proprio per disporre di un quadro maggiormente aggiornato della situazione, il prefetto ha convocato una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la sede del palazzo municipale di Carovigno. In tale circostanza, da un lato, è stato dato impulso a mirati servizi delle forze di polizia nell'ambito del piano coordinato di controllo del territorio, dall'altro, in un'ottica di sicurezza partecipata, non si è mancato di incentivare la collaborazione della polizia municipale. A tale proposito, informo che l'amministrazione comunale per il periodo estivo ha assicurato il proprio impegno nel promuovere misure organizzative volte ad incrementare le unità di polizia locale con assunzioni a tempo determinato, anche allo scopo di liberare risorse che possano concorrere, nell'ambito delle proprie competenze, al controllo coordinato del territorio. Quanto alla presenza delle Forze dell'ordine sul territorio comunale, la stazione dei carabinieri di Carovigno registra un organico effettivo di dodici unità, ritenuto adeguato alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica dei territorio, anche perché il rapporto carabinieri-abitanti risulta in linea con il dato nazionale e più favorevole rispetto al dato regionale. Su un piano più generale, rappresento per completezza che il complessivo dispositivo di sicurezza presente a livello provinciale si compone di 1.651 unità di personale, di cui 512 unità appartenenti alla Polizia di Stato, 538 militari dell'Arma dei carabinieri e 601 unità di personale appartenente alla Guardia di finanza. Per quel che concerne infine le dotazioni tecnologiche in materia di videosorveglianza, rilevo che tutta la zona del centro storico del Comune in questione è stata dotata di un sistema di videosorveglianza finanziato di recente con fondi del precedente Programma operativo nazionale sicurezza. Vi è l'intendimento, previo reperimento di ulteriori finanziamenti, di implementare il dispositivo con l'installazione, anche nelle zone di accesso al paese, di ulteriori punti di videosorveglianza che, oltre a costituire un deterrente, sono ovviamente un valido supporto per l'attività investigativa delle Forze dell'ordine. Assicuro, in conclusione, che la situazione della sicurezza e dell'ordine pubblico a Carovigno è continuamente monitorata anche da parte del Ministero Ministero ed è oggetto di costante attenzione da parte delle autorità provinciali di pubblica sicurezza e delle forze di polizia, che non mancheranno di adottare, all'occorrenza, ogni opportuna misura diretta a rendere ancora più efficaci gli attuali dispositivi di controllo del territorio.

questi militari siano impegnati anche in tali servizi. Quindi, chiedo se il Governo possa valutare, anche in base a queste nuove esigenze, la possibilità

e soprattutto per le tante persone che lavorano nel settore, non avere l'opportunità di dare sicurezza ai turisti che sono ormai fonte di reddito importante per tutti noi.

all'ordine del giorno il senatore Crimi richiede una serie di dati relativi al fenomeno dei suicidi tra gli appartenenti alle Forze di polizia e alla polizia municipale, con riferimento al periodo compreso tra il 2009 e il 2014. Per quanto concerne la Polizia di Stato, nel periodo in esame, si sono registrati 62 suicidi, di cui tre hanno riguardato personale di sesso femminile. L'età media dei soggetti coinvolti è di quarantaquattro anni. Per quanto riguarda le modalità, in 50 casi è stata utilizzata la pistola di ordinanza, in quattro casi un altro tipo di arma, mentre i restanti otto eventi hanno avuto corso con altre dinamiche. Quanto all'Arma dei carabinieri, nello stesso periodo di riferimento, si sono registrati 92 eventi, di cui solo uno ha riguardato una donna. L'arma da fuoco è stata utilizzata in 80 casi. L'età media dei soggetti coinvolti oscilla tra i circa trentanove anni nel 2014 Il dato riferito alla Guardia di finanza è di 45 casi di suicidio riguardanti solo personale di sesso maschile, con un'età media di circa In 41 casi è stata utilizzata l'arma di ordinanza, in 4 casi l'evento si è verificato con modalità diverse. Nel Corpo di polizia penitenziaria si sono registrati 47 eventi, tutti riguardanti personale di sesso maschile. In merito alle modalità, 30 suicidi sono avvenuti con arma di ordinanza e due con arma personale, mentre gli altri 15 casi hanno avuto dinamiche diverse. L'età media dei soggetti coinvolti è di circa Con riferimento al Corpo forestale dello Stato, sono stati accertati otto suicidi, di cui sei hanno riguardato uomini e due donne, tutti eseguiti con l'arma di ordinanza. L'età media dei soggetti coinvolti è ancora una volta di Riferisco, infine, che il Ministero dell'interno non dispone di dati relativi all'incidenza del fenomeno nei Corpi di polizia locale, perché tali dati non affluiscono al Ministero dell'interno. Ai fini di una corretta lettura dei dati che ho appena fornito, preme evidenziare che il miglioramento delle condizioni lavorative e di vita del personale delle forze di polizia è uno degli obiettivi prioritari dei Dicasteri di rispettiva appartenenza. Per quanto Per quanto riguarda questa Amministrazione, segnalo, a dimostrazione dell'attenzione riservata al tema, che da diversi anni la Direzione centrale di sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza ha attivato numerose iniziative in materia di prevenzione e gestione del disagio psichico nel personale della Polizia di Stato e di sostegno in occasione di eventi critici e ad alto impatto emotivo anche non inerenti ad attività di servizio. In tale ambito, la predetta Direzione centrale, anche avvalendosi della collaborazione di docenti universitari ed esperti del settore, monitora e analizza costantemente il fenomeno. L'esame dei dati acquisiti non evidenzia un incremento numerico dei suicidi, ma un andamento discontinuo, mentre la valutazione delle singole fattispecie esclude che gli eventi in parola siano riconducibili a problematiche di disagio lavorativo o comunque a situazioni critiche connesse all'attività svolta. Rappresento, inoltre, che è in fase di elaborazione un documento, frutto di uno studio sistematico di tale problematica, che fornirà tutti i dati di dettaglio ed individuerà ulteriori iniziative tese alla prevenzione del fenomeno nell'ambito della Polizia di Stato. Le risultanze preliminari di questo studio non forniscono - almeno allo stato - elementi di allarme. Infine, il Ministero della giustizia ha tenuto a precisare che al tema del benessere del personale della Polizia penitenziaria è stato dedicato un apposito spazio nel contesto dell'articolata iniziativa degli Stati generali sull'esecuzione penale; benessere da realizzarsi attraverso il potenziamento della sorveglianza dinamica e la valorizzazione del personale e della sua formazione. Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario perché finalmente dopo più di un anno riusciamo ad avere questi dati: erano dei numeri. Tendenzialmente quella era la richiesta dell'interrogazione; non si chiedeva altro, semplicemente dei numeri che è difficile reperire. Ci sono delle associazioni che fanno degli sforzi immani, si affidano a dati pubblici - quelli che trovano sulla stampa - per poter raccogliere queste informazioni e poter capire qualcosa di più. Non è però soddisfacente il fatto che sia la stessa amministrazione a cercare le eventuali cause o connessioni. Rendere pubblici i dati, renderli disponibili anche all'esterno, a ricercatori o altri soggetti che possono svolgere approfondimenti, fa sì che il risultato possa essere più oggettivo. Infatti, che lei mi dica che non c'è una correlazione

c'è uno stress accumulato e a volte non è possibile identificare situazioni di stress o criticità legate a eventi che all'apparenza possono sembrare ordinari. Basti immaginare un agente della polizia locale o della polizia stradale che deve intervenire in un incidente stradale in cui una delle vittime è un bambino di età simile a quella di un suo figlio che All'apparenza sembra un intervento ordinario, ma immaginate quale può essere la conseguenza emotiva per quella persona e cosa si porta a casa, dove poi trova suo figlio, e cosa può succedere.

tentativi hanno tutti questa fine tragica. Crediamo inoltre che non sia sufficiente il supporto psicologico interno. Anche questo è un altro elemento che bisognerebbe andare ad approfondire. Non si può sovrapporre la figura del valutatore con quella di chi fa supporto psicologico, perché sappiamo bene che quando si va a denunciare uno stato d'animo, uno stato emotivo che può avere una causa scatenante per effetti tragici,

si valuta se sia avvenuto a seguito di un evento critico specifico, dimenticando che i soggetti che compiono questo gesto spesso sono al termine di un processo di decadimento. È vero che i suicidi sono tra i

Signor Presidente, con l'interrogazione all'ordine del giorno il senatore Davico, nel richiamare le vicende che hanno portato all'annullamento parziale delle elezioni amministrative per la carica di sindaco di Voghera del maggio-giugno 2015, solleva perplessità sull'operato del commissario prefettizio posto provvisoriamente a capo dell'amministrazione comunale, con particolare riferimento alla nomina dei vertici della società partecipata ASM Voghera SpA. Prima di esaminare le questioni poste dall'interrogante, ritengo necessario soffermarmi brevemente sulle vicende che hanno condotto il prefetto di Pavia a nominare il citato commissario; vicende richiamate con qualche accenno critico nel preambolo dell'atto di sindacato ispettivo. Al turno di ballottaggio elettorale, tenutosi il 14 giugno 2015, Carlo Barbieri ha riportato più voti dell'altro candidato ammesso al secondo turno, Aurelio Torriani, ed è stato confermato quindi

sindaco, Pier Ezio Ghezzi, escluso dal ballottaggio per uno scarto di quattro voti rispetto ad Aurelio Torriani. In sede di esame del ricorso, il TAR ha incaricato la prefettura di Pavia di procedere «in contraddittorio con le parti, debitamente avvisate, alla verificazione dei voti totali conseguiti dai candidati Ghezzi e Torriani» limitatamente a due sezioni elettorali. Le operazioni svolte dalla commissione istituita *ad hoc* dal prefetto, composta da tre membri tra i quali il vice prefetto Sergio Pomponio, hanno evidenziato una discrepanza dei risultati finali rispetto ai numeri riportati nei verbali delle predette sezioni, ribaltando l'esito delle elezioni comunali del 31 maggio 2015 in senso favorevole al ricorrente. La bontà dell'operato della commissione prefettizia è stata riconosciuta dal TAR per la Lombardia che, con sentenza del 17 febbraio scorso, ha accolto il ricorso del candidato sindaco Pier Ezio Ghezzi. Il medesimo provvedimento giurisdizionale, inoltre, nella motivazione, ha evidenziato che «l'annullamento della competizione elettorale, seppure in parte, determina l'automatica cessazione delle funzioni del sindaco sindaco attualmente in carica, spettando all'Autorità prefettizia le determinazioni in ordine al governo dell'ente nella fase precedente la conclusione della procedura di ripetizione del turno di ballottaggio». Più di recente, il 21 luglio scorso, il Consiglio di Stato, oltre a confermare la correttezza dell'operato della Prefettura nella decisione di procedere allo scioglimento del Consiglio comunale, ha respinto l'appello proposto dal sindaco uscente Carlo Barbieri. In ottemperanza alle statuizioni del TAR Lombardia, il prefetto di Pavia ha sospeso gli organi elettivi del Comune di Voghera, nominando il vice prefetto Sergio Pomponio commissario prefettizio dell'ente fino alla conclusione della procedura di ripetizione del turno di ballottaggio. La scelta è caduta sul dottor Pomponio sia in ragione dei rilevanti incarichi ricoperti nella prefettura, cioè vice prefetto vicario e dirigente reggente dell'area preposta ai rapporti con gli enti locali, sia per l'esperienza maturata nelle gestioni commissariali, avendo il predetto già ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di subcommissario dei Comuni di Parma e di Venezia. Vengo ora alle doglianze del senatore Davico circa il procedimento di nomina del consiglio di amministrazione della società partecipata ASM Voghera SpA; doglianze riferite, in particolare, alla nomina della dottoressa Barbara Piermarioli alla carica di presidente dell'organismo. Mi corre l'obbligo di riferire anzitutto che l'ordinamento vigente non conferisce né ai prefetti titolari di sede provinciale, né ad altri organi del Ministero dell'interno poteri di controllo di legittimità degli atti dei Comuni. Ciò vale anche nelle ipotesi in cui l'ente locale è retto provvisoriamente da un commissario di nomina prefettizia o presidenziale. Tanto premesso, in ordine agli specifici quesiti posti dal senatore interrogante sul nuovo consiglio di amministrazione della società partecipata ASM Voghera, il commissario Pomponio ha fornito alla prefettura di Pavia le informazioni che si riportano sinteticamente di seguito. Il rinnovo del consiglio di amministrazione si è reso necessario, ai sensi dello statuto di quell'ente, a seguito alle dimissioni presentate nello scorso mese di febbraio da tre dei cinque consiglieri. Nel procedere a tale adempimento, il dottor Pomponio ha preso preliminarmente atto che gli indirizzi e i criteri dettati dal Consiglio comunale di Voghera per le nomine e le designazioni di competenza del Sindaco si adattano solo in parte alla figura del commissario prefettizio, caratterizzata dalla monocraticità dei poteri e dall'assoluta provvisorietà e indeterminatezza temporale dell'incarico. Quindi, ha ritenuto necessario far precedere la nomina del consiglio di amministrazione della ASM Voghera da un atto di indirizzo *ad hoc*, pubblicato all'albo pretorio *online* e quindi facilmente e tempestivamente consultabile da In tale documento il commissario, oltre a prevedere la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione da cinque a tre, in coerenza con i principi posti dalla più recente normativa in tema di riordino delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, ha reso noti i criteri generali a cui si sarebbe attenuto nella nomina dell'organismo collegiale in questione: dare dare alla ASM Voghera una conduzione di profilo prettamente tecnico, in grado di assicurare la piena efficienza e funzionalità dell'azienda nella delicata fase di recepimento delle importanti novità introdotte dal legislatore nel settore; procedere a nomine di professionisti legati da un rapporto strettamente fiduciario con il commissario prefettizio medesimo; applicare rigorosamente il principio secondo il quale gli organi di amministrazione elettiva del Comune di Voghera, in atto sospesi, possano riassumere integralmente, al termine della gestione commissariale, senza ostacolo o condizionamento alcuno, il potere/dovere di effettuare ogni valutazione e decidere le scelte strategiche in merito alle prospettive della società, nominando un consiglio di amministrazione di propria diretta espressione. Sulla base dell'atto d'indirizzo, adottato il 29 marzo scorso con i poteri della Giunta e con dovizia di motivazioni circa ciascuna delle scelte compiute, nella stessa giornata il commissario ha nominato - stavolta con i poteri del sindaco - il nuovo consiglio di amministrazione, conferendo le funzioni di presidente alla dottoressa Piermarioli. Ricostruita così la vicenda, il commissario prefettizio ha inteso ribadire la correttezza del proprio operato complessivo, confutando anche alcuni specifici rilievi critici contenuti nell'interrogazione. Quanto alle circostanze di non aver attinto, per le nomine in questione, alle candidature presentate quando gli organi comunali elettivi erano ancora operanti e di non aver riaperto i termini per la presentazione di nuove candidature, il commissario prefettizio ha precisato di non aver seguito tali strade non per un giudizio aprioristico di demerito o incompetenza professionale delle persone candidate, ma perché si sarebbe trattato di soluzioni non adeguate in relazione alla peculiarità della gestione commissariale. Circa l'affermazione che i consiglieri di amministrazione nominati sono «estranei alla città», con la conseguenza che ciò comporta «notevoli ed inevitabili spese di trasferta», il commissario ha precisato che i rimborsi sono consentiti dalla legge e avverranno comunque nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la materia; d'altro canto, ha invitato a considerare positivamente la circostanza che i compensi fissi e variabili dei neopresidente e vicepresidente della ASM Voghera sono individualmente inferiori, in maniera significativa, a quelli previsti fino al 2015 per le analoghe cariche cessate. Sotto i diversi profili della correttezza istituzionale e della trasparenza amministrativa, un altro aspetto sicuramente da apprezzare è l'impegno assunto dai nuovi amministratori di cessare dall'incarico al termine del mandato del commissario, ovviamente in linea con una delle precisazioni iniziali fatta dallo stesso commissario. Per quanto riguarda la nomina della dottoressa Piermarioli a presidente della società in questione, sempre il dottor Pomponio ha rappresentato che la scelta è stata dettata dal *curriculum* di tutto rispetto della professionista, che vanta al suo attivo significative esperienze di amministratrice di società pubbliche, revisore dei conti, curatrice fallimentare, consulente tecnica, *advisor* per la predisposizione di piani concordatari concordatari e commissaria giudiziale di aziende, senza trascurare la collaborazione quindicennale con il tribunale di Parma. Con riferimento al procedimento penale avviato dalla procura della Repubblica di Parma a carico della dottoressa Piermarioli, si sottolinea che le cause di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi negli enti pubblici, nelle aziende e nelle società a totale o parziale capitale pubblico sono stabilite dalla legge in modo tassativo e al momento nessuna di esse risulta ricorrere nei confronti della predetta professionista. Tra l'altro, agli atti del Comune è depositata una dichiarazione resa in tal senso dall'interessata all'atto di accettazione della nomina a Presidente della ASM Voghera.

Di fatto bisogna fare molta attenzione perché si tratta del momento più importante della democrazia e della partecipazione dei cittadini. In secondo luogo, quando gli organi dello Stato interagiscono tra di loro per queste vicende,

questi aspetti non stati rispettati, non sono stati osservati e quindi si è intervenuti in modo non corretto o se non altro inopportuno e indelicato dal punto di vista di quella attenzione e di quella presenza che noi dovremmo manifestare attraverso soggetti come il Ministro dell'interno che sono preposti a simili interventi. Intanto c'è una inopportunità nella tempistica: questa interrogazione è di aprile, sono passati mesi e qui abbiamo una democrazia sospesa: bisogna darsi da fare subito, bisogna intervenire subito, bisogna rispondere subito

ancora l'inopportunità nella nomina di quel commissario, ma non per la persona, perché non ci interessano qui le persone. Chi rifà il conteggio probabilmente, per un'opportunità democratica, non dovrebbe essere quello che poi fa il commissario.

l'evoluzione del fatto democratico, del fatto elettorale e, dunque, la conclusione più positiva possibile delle vicende.

ad un avviso di garanzia emesso dalla procura della Repubblica di Caltagirone nei confronti di sei persone coinvolte a vario titolo nella gestione del CARA di Mineo. Prendendo spunto da tale vicenda, la senatrice pone una serie di quesiti volti a conoscere quali misure il Ministero dell'interno intenda adottare in relazione alla preoccupante situazione di illegalità che sarebbe emersa dalle indagini. Secondo quanto riferito dal Ministero della giustizia, appositamente interpellato sul procedimento penale in questione, gli accertamenti della predetta procura hanno evidenziato che, nel periodo compreso tra l'ottobre 2011 e il giugno 2015, sarebbero state rendicontate spese di gestione relative a migliaia di ospiti dimessi e cancellati formalmente dal CARA di Mineo in data successiva a quella del loro effettivo allontanamento dal centro, con conseguente erogazione da parte dello Stato italiano e, in misura minore, da parte dell'Unione europea, di somme non dovute per un ammontare complessivo di poco superiore ad un milione di euro. In relazione a tale condotta, la procura di Caltagirone ha notificato un decreto di perquisizione e sequestro e contestuale informazione di garanzia alle sei persone citate nel testo dell'interrogazione, contestando loro i reati di falsità ideologica e truffa aggravata, commessi in tempi diversi, in concorso e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, Al riguardo, voglio subito sottolineare che i fatti oggetto di accertamento penale risalgono a un'epoca in cui nessun organo del Ministero dell'interno ha svolto, in relazione alla struttura di Mineo, ruoli o attività specifiche che riguardassero aspetti contrattuali o gestori o che comunque fossero ricollegati alla scelta degli affidatari. In effetti, nel quinquennio 2011-2015, tali compiti sono stati svolti, con diversi livelli di responsabilità, dal Consorzio dei comuni «Calatino terra di accoglienza» e da un'associazione temporanea di imprese sulla base di un contratto di appalto stipulato tra gli stessi. Fatta questa doverosa premessa, al fine di rispondere ai quesiti posti dagli interroganti e alla domanda di legalità e trasparenza che essi sottendono, ritengo opportuno ripercorrere le azioni e i provvedimenti adottati adottati dal sistema Stato per superare le criticità emerse nella gestione del CARA di Mineo. Quando dico «sistema Stato», faccio riferimento principalmente all'azione della magistratura, dell'Autorità nazionale anticorruzione e ovviamente del Ministero dell'interno. Il 4 giugno 2015 è stata eseguita, nell'ambito del procedimento penale sul sodalizio Mafia Capitale, l'ordinanza del gip presso il tribunale di Roma che ha disposto misure cautelari anche nei confronti del Consorzio di cooperative sociali Casa della Solidarietà La Cascina Global Service Srl, facenti parte dell'associazione temporanea di imprese, di cui parlavo prima, aggiudicataria dei servizi di gestione della struttura di Mineo. Nell'occasione, la magistratura inquirente ha contestato la presunta commissione dei reati di corruzione e di turbata libertà degli incanti. Dall'esame dell'ordinanza cautelare, l'ANAC ha rilevato la sussistenza di accordi corruttivi e condotte fraudolente tali da concretare gli estremi per il commissariamento delle predette società, ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014.

Le due società sono state destinatarie anche di un provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla prefettura di Roma il giorno precedente, cioè il 22 giugno, nonché della misura di prevenzione patrimoniale dell'amministrazione giudiziaria decretata il 27 luglio dal tribunale capitolino, ai sensi del codice antimafia. In relazione a quest'ultima misura, il 10 agosto, il prefetto di Catania, d'intesa con l'Autorità anticorruzione, ha adottato un provvedimento di sospensione del commissariamento precedentemente disposto ai sensi del decreto-legge n. 90 del 2014. Sempre nel 2015, si è registrato un altro importante sviluppo. Il 23 novembre, la prefettura di Catania, su indicazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è subentrata al Consorzio dei comuni «Calatino terra di accoglienza» nei rapporti contrattuali con l'associazione temporanea di imprese preposta alla gestione della struttura di Mineo. In considerazione della complessità degli adempimenti da svolgere, la prefettura è stata affiancata da una struttura di missione *ad hoc* composta da due dirigenti della carriera prefettizia e da sei unità di personale non dirigenziale, con importanti compiti di controllo e monitoraggio, oltreché di preparazione della procedura di gara per la scelta da parte della prefettura medesima del nuovo soggetto gestore del CARA di Mineo. Tra tali compiti si annovera anche la verifica di congruità delle fatture emesse dall'associazione temporanea di imprese e trasmesse periodicamente alla prefettura di Catania. La verifica viene effettuata riscontrando il registro delle presenze degli ospiti del centro con le relative movimentazioni in entrata e in uscita. All'ingresso del centro è stato collocato un sistema di rilevazione automatica delle presenze che, attraverso un apposito tesserino magnetico di riconoscimento, registra le entrate e le uscite di ciascun ospite. È prevista anche la disattivazione automatica dei *badge* non utilizzati per tre giorni consecutivi. Il pagamento delle fatture viene effettuato successivamente dalla prefettura sulla base della verifica di congruità e dei controlli ordinari eseguiti dalla struttura di supporto sulla documentazione contabile del CARA. Ritengo che la ricostruzione dei fatti appena esposta evidenzi come, nel giro di poco più di un anno, oltre ad avviare l'avvicendamento dei soggetti gestori del centro di Mineo, siano state introdotte nuove ed incisive procedure gestionali e di controllo miranti, proprio nel senso auspicato dagli interroganti, a prevenire episodi di illegalità come quelli scoperti e perseguiti dalla procura della Repubblica di Caltagirone. Ciò costituisce la conferma che il Ministero dell'interno è organo perfettamente interessato e garante della trasparenza e della legalità, come dimostrato anche dal ruolo giocato dal prefetto di Catania, oltre che da quello di Roma. Questa amministrazione ha dunque tutto l'interesse a che la struttura di Mineo operi secondo una nuova prospettiva fondata sulla riconsiderazione del sistema di affidamento e dei meccanismi di gestione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza. Concludendo, informo, per completezza, che nello scorso mese di luglio il prefetto di Catania, preso atto della cessazione dell'amministrazione giudiziaria dei due dei soggetti gestori del CARA di Mineo ad opera del tribunale di Roma, ne ha disposto nuovamente la sottoposizione alla gestione straordinaria e temporanea, ai sensi del decreto-legge 11 agosto 2014, n. 90. Infine, con riferimento al nuovo CARA di Mineo, struttura più volte menzionata nel testo dell'interrogazione, la prefettura di Catania ha fatto sapere che si tratta di un consorzio di scopo che l'associazione temporanea di imprese che gestisce il CARA di Mineo ha istituito al proprio interno per una migliore organizzazione dei servizi di assistenza alle persone. Con tale consorzio la prefettura non ha mai intrattenuto alcun rapporto diretto, neanche di natura contrattuale.

nonostante lei mi stia dicendo che la prefettura non ha alcun contatto diretto con queste persone, con la nostra interrogazione presentata qualche mese fa volevamo sollecitare la vostra attenzione proprio su questo.

riscontriamo puntualmente che quanto scritto negli organigrammi e nel programma di gestione delle persone a livello umano, educativo e di inserimento non corrisponde mai a quello che realmente si realizza. Quando si parla di minori, è chiaro che la situazione si aggrava. In ogni caso, a nostro avviso, rimane il quesito su questa *task force* ispettiva che il Governo intende

hanno fatto dei video e un *reportage* molto dettagliato sulle condizioni veramente raccapriccianti di vita dei migranti. A nostro avviso, non bisogna lasciare questo tema inosservato, anche se avete fatto dei passi avanti e istituito questi *budget* che sicuramente possono

Signora Presidente, mediante l'atto ispettivo in oggetto, gli onorevoli interroganti ripercorrono la vicenda giudiziaria relativa al magistrato Giuseppe Recupero che, in qualità di presidente della corte d'assise di Messina, aveva emesso sentenza di assoluzione nei confronti dei fratelli Michele e Salvatore Greco in ordine alla imputazione di concorso nell'omicidio del consigliere istruttore Rocco Chinnici, e che era stato, successivamente, indagato dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria per concorso esterno in associazione mafiosa ed altro. Evidenziano, in particolare, come in seguito alla declinazione di competenza del giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria, in data 7 luglio 1998, il fascicolo processuale fosse stato trasmesso alla procura della Repubblica di Palermo, dove, tuttavia, lo stesso non veniva iscritto nel registro generale delle notizie di reato sino al 2013, quando si era dato corso agli adempimenti conseguenti al provvedimento di trasmissione ed il procedimento era stato archiviato per essere l'indagato ormai deceduto. Censurano, pertanto, l'inerzia della procura palermitana che, per ben quindici anni, non avrebbe provveduto all'iscrizione ed agli adempimenti conseguenti, chiedendo se il Ministro della giustizia sia a conoscenza dei fatti e quali iniziative intenda assumere per l'accertamento delle relative responsabilità. Quanto alla ricostruzione della vicenda processuale esposta, si riporta testualmente la nota trasmessa dal procuratore della Repubblica di Palermo, nella quale si legge come il predetto ufficio «ebbe a ricevere nel 1998 dall'autorità giudiziaria di Reggio Calabria due distinti procedimenti, facenti parte però di un unico filone di indagini: il primo, trasmesso dal tribunale di Reggio Calabria a seguito di sentenza di incompetenza emessa da quel gup (pronunciata il 21 maggio 1998),

il secondo, trasmesso dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria a seguito di ordinanza dichiarativa di incompetenza emessa dal gip della stessa sede (in data 4 marzo 1998), venne inviato parzialmente in copia dalla procura di Reggio Calabria e ricevuto da quest'ufficio il 14 14 luglio 1998 (nella nota di trasmissione, il pubblico ministero di Reggio Calabria evidenziava che l'intero fascicolo in originale, inclusa quindi la parte definita con sentenza, era stato già trasmesso dall'ufficio del successivamente, altri atti riguardanti il Recupero Giuseppe e Scarpisi Pietro pervennero a quest'ufficio in data 8 agosto 1998». Aggiunge il procuratore che soltanto il secondo di detti procedimenti, nei confronti di cinque soggetti, venne iscritto al registro notizie di reato di quest'ufficio e si concluse con richiesta di archiviazione del 20 agosto 1998, accolta dal gip presso il tribunale di Palermo in data 11 settembre 1998. Nessuna iscrizione risulta invece effettuata - ma sul punto il procuratore formula riserva di elementi aggiuntivi in attesa del completamento delle verifiche con riferimento al procedimento proveniente dal tribunale di Reggio Calabria, nei confronti di Recupero Giuseppe e Scarpisi Pietro. Gli atti del relativo procedimento risultavano in qualche modo inseriti nell'unico fascicolo oggetto anche dell'ordinanza di incompetenza. Detto procedimento venne invero rinvenuto soltanto nel 2013. Il procuratore della Repubblica ne dispose l'iscrizione nel registro modello 21, provvedendo alla sua assegnazione. Detto procedimento è stato poi definito con richiesta di archiviazione anche nel merito con riferimento alla posizione dello Scarpisi che parzialmente refluisce su quella del Recupero, frattanto deceduto, in data 25 novembre 2013, pienamente e *de plano* accolta dal gip di Palermo in data 6 dicembre 2013. L'*iter* procedimentale è stato, pertanto, circostanziato nei termini riportati dalla competente procura. Quanto all'esercizio delle prerogative riconosciute al Guardasigilli secondo la Costituzione e le leggi, ogni opportuna valutazione in merito verrà svolta dal Ministro della giustizia all'esito della trasmissione, da parte del procuratore della Repubblica di Palermo, dei risultati dell'attività di verifica di cui ha fatto riserva. In attesa degli esiti degli accertamenti, pertanto, si rassicurano gli onorevoli interroganti della massima attenzione che il Ministro riserverà, nell'ambito delle proprie attribuzioni, alla vicenda, tenendo in debita considerazione anche la sua delicatezza e particolare complessità.

rimanga in piedi un'ipotesi accusatoria gravissima a carico di un magistrato, un presidente di sezione, accusato di avere percepito 200 milioni di lire e addirittura un cavallo da parte delle cosche

E stiamo parlando di dare giustizia a un servitore dello Stato, Rocco Chinnici, ai carabinieri che lo scortavano,

chi aveva il compito di dirci se quel magistrato fosse o no colpevole di quanto era accusato. E noi le ricordiamo quelle vicende. quelle vicende. Quel processo veniva da due decisioni delle corti di merito di condanna dei fratelli Greco, entrambe annullate in Cassazione di mafiosi annullate da Corrado Carnevale. La sentenza che condanna i mandanti della strage Chinnici dice che non si possono condannare i Greco, perché è passato il giudicato: quel vergognoso giudicato.

Alcuni addirittura ignoti, come dice la sentenza, e altri ricoperti dal giudicato. Vergognoso! Quindi, signora Sottosegretaria, noi non possiamo sentirci soddisfatti da questa risposta, a distanza di così tanto tempo.

mediante l'atto di sindacato ispettivo in discussione - che richiama una nota, riportata dalla stampa, indirizzata dal procuratore della Repubblica di Bari al Ministero della giustizia per rappresentare la situazione di criticità in cui versa l'ufficio della procura distrettuale di Bari per la carenza di personale amministrativo si chiede di conoscere quali iniziative, di tipo normativo ed organizzativo, il Ministro intenda adottare al fine di garantire *standard* minimi di funzionamento del sistema giudiziario. In riferimento alle specifiche questioni prospettate, si ribadisce, anche in questa sede, che l'adozione di strutturali misure a sostegno degli uffici giudiziari ha costituito obiettivo prioritario dell'azione del Ministro della giustizia, perseguito - tra l'altro - attraverso nuove politiche per il personale amministrativo negli uffici giudiziari, dopo anni di assoluta stagnazione. Dalle informazioni trasmesse dalla competente articolazione ministeriale, risulta che presso la procura della Repubblica di Bari risultano attualmente in servizio 123 unità di personale amministrativo rispetto alla previsione, in pianta organica, di 134 risorse umane, con una percentuale di scopertura dell'8,21 per cento, inferiore alla media nazionale del 21,80 Nello specifico, con particolare riferimento ai profili di maggior rilievo, ai fini del corretto funzionamento dell'ufficio, risulta che la posizione dirigenziale è temporaneamente coperta mediante reggenza e che sono interamente completi gli organici del funzionario contabile, dell'operatore giudiziario, del conducente di automezzi e dell'ausiliario. Quanto ai funzionari giudiziari, un posto già vacante è stato coperto con uno dei vincitori del bando di mobilità esterna pubblicato nel 2015. In seguito alla procedura di interpello per i trasferimenti a domanda del personale dell'amministrazione giudiziaria sono stati, inoltre, coperti entrambi i posti pubblicati (uno di funzionario giudiziario ed uno di funzionario contabile), mentre è uscita dall'ufficio una sola unità (un cancelliere). All'esito della prima fase della procedura di mobilità obbligatoria, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, gestita attraverso il portale della funzione pubblica, è stato, inoltre, assunto un direttore amministrativo, proveniente dagli elenchi di personale in esubero, che ha assunto possesso nell'ufficio lo scorso 1° settembre. Con le procedure di acquisizione del personale posto in mobilità obbligatoria, hanno preso complessivamente servizio il 1° settembre scorso, sul territorio nazionale, 344 nuove risorse di personale, di cui 73 provenienti dagli enti di area vasta e 286 da altri settori. L'equiparazione delle loro mansioni e profili è avvenuta ai sensi della normativa vigente, ma il Ministero ha già programmato specifici percorsi di formazione. Ulteriori unità potranno essere reclutate una volta completate le procedure di mobilità obbligatoria e, contestualmente allo sblocco del *turnover*, sarà inoltre possibile riprendere le ordinarie capacità assunzionali. Uno specifico emendamento al decreto-legge sul processo amministrativo telematico, convertito con legge approvata dal Parlamento il 3 agosto scorso, prevede ora l'assunzione a tempo indeterminato di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale nel Ministero della giustizia. La legge prevede, inoltre, la possibilità di introdurre nuovi profili professionali, anche tecnici, fondamentali per la gestione delle spese di funzionamento degli uffici e la digitalizzazione avanzata. Proprio per dare attuazione ad un quadro normativo che ha avviato straordinarie procedure di reclutamento di nuove risorse attraverso bandi di mobilità volontaria, mobilità obbligatoria, riqualificazione e, infine, nuove assunzioni grazie al decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, che non solo autorizza il Ministero ad un vero e proprio programma assunzionale, ma completa efficacemente un complessivo quadro di disposizioni legislative in materia di personale, il Guardasigilli ha indirizzato, lo scorso 8 settembre, ai capi degli uffici una direttiva contenente le linee di intervento a cui far riferimento. La direttiva intende assicurare al nuovo personale la più idonea e adeguata formazione, valorizzando le competenze già diffuse nei vari uffici sul territorio e facendo ricorso a più innovativi ed agili strumenti di formazione. Saranno, inoltre, rivisti e rimodulati i profili professionali, riconsiderata la definizione di alcune mansioni e inserite nuove figure professionali, attualmente non presenti nell'amministrazione della giustizia, secondo un piano di linee di intervento che completa efficacemente il complessivo quadro di disposizioni legislative in materia di personale già avviato. Nell'ambito dell'articolato programma di nuove assunzioni per la giustizia che si sta in tal modo delineando, anche all'ufficio in disamina potranno essere assegnate nuove risorse. Analogo impegno è stato profuso per assicurare agli uffici adeguate dotazioni di personale di magistratura. In questa prospettiva, l'assetto conseguente alla riforma della geografia giudiziaria è stato oggetto di continua osservazione, nel complesso degli interventi, non ancora esauriti, di tipo normativo e organizzativo, necessari a costruire una struttura ordinamentale idonea a rispondere in modo soddisfacente alla domanda di giustizia e alle esigenze del territorio. percorso di revisione sta ora attraversando una ulteriore, importante fase, con l'invio al Consiglio superiore della magistratura dello schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado, conseguente proprio alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, e che recepisce le esigenze degli uffici secondo la loro dislocazione territoriale. In tale contesto, è stato previsto l'aumento dell'organico della procura della Repubblica di Bari di un posto di procuratore aggiunto e di due posti di sostituto procuratore. Preme evidenziare che l'aumento di un posto di procuratore aggiunto risponde alle finalità proprie delle procure distrettuali antimafia, mirando ad assicurare una maggiore efficacia all'azione di contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, nel caso di specie particolarmente gravi ed allarmanti nel circondario di Foggia. Quanto alla determinazione delle unità aggiuntive, la stessa è stata effettuata sulla base di parametri statistici - popolazione, flussi, *cluster* dimensionali integrati da indicatori qualificativi della domanda di giustizia, quali il numero di imprese presenti sul territorio e la loro concentrazione per circondario, l'incidenza della criminalità organizzata, l'accessibilità del servizio per i cittadini (i cosiddetti *city user*). Alla stregua della lettura combinata dei predetti indicatori, pertanto, la procura della Repubblica di Bari è stata dotata di unità aggiuntive, nel più ampio incremento del personale di magistratura del distretto, che vede complessivamente assegnati agli uffici giudiziari baresi sette posti di giudice e due di sostituto procuratore della Repubblica. Quanto, invece, alle iniziative finalizzate a modificare le misure del codice penale adottate in tema di improcedibilità per tenuità del fatto e di depenalizzazione di talune fattispecie, allo scopo di garantire il buon funzionamento del servizio giustizia - pure prospettate nell'interrogazione - si rappresenta come non siano allo studio ulteriori iniziative normative in materia, in considerazione della recente entrata in vigore degli istituti deflattivi. Per ovviare ad eventuali criticità o problemi interpretativi derivanti dalla applicazione del nuovo testo normativo, la stessa legge delega ha previsto, peraltro, la possibilità di emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di attuazione, uno o più decreti correttivi ed integrativi. Il che lascia aperta la strada normativa per eventuali correttivi, ritenuti necessari all'esito dei primi monitoraggi svolti.

prendendo a base i dati risultanti dal monitoraggio degli effetti dell'intervento normativo ai fini di eventuali modifiche correttive. Con specifico riferimento, infine, a quanto dedotto nell'atto ispettivo in ordine alla possibilità di destinare parte delle risorse che confluiscono nel Fondo unico di giustizia (FUG) al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari (tra cui, nella specie, quelli della Procura della Repubblica barese) si rappresenta che - come noto - l'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge n. 181 del 13 novembre 2008, ha affidato ad Equitalia Giustizia SpA la gestione del Fondo. In ordine alla distribuzione delle risorse confluite nel FUG, l'articolo 2, del 2008 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, sono stabilite le quote delle risorse disponibili da destinare, mediante riassegnazione, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia, oltre che al bilancio dello Stato. Il regolamento di attuazione n. 127 del 2009 stabilisce, poi, all'articolo 7, che l'immediata riassegnazione delle somme ai Ministeri della giustizia e dell'interno è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti sinora emanati hanno sempre previsto la destinazione del 49 per cento al Ministero dell'interno, del 49 per cento al Ministero della giustizia e del 2 per cento al bilancio dello Stato. Negli anni 2011-2015 il Ministero della giustizia ha conseguito, a titolo di anticipazione, la somma complessiva di 600.520.000 euro. L'ammontare delle risorse destinate al Ministero della giustizia è pertanto determinato dai vigenti parametri normativi.

apprezzo lo sforzo con cui si è tentato di dare una risposta alla mia interrogazione, risposta che considero assolutamente insufficiente, perché sostanzialmente non si offre, neanche in termini di prospettiva, una soluzione alle complesse

ha portato a conoscenza del signor Ministro guardasigilli. Per quanto attiene all'ultimo punto evidenziato, concernente il Fondo unico della giustizia, si è quantizzata la somma che in quota parte è stata assegnata al Ministero della giustizia, ma non si dà una risposta in ordine a quale somma di questo Fondo è stata destinata, così come previsto e ricordato peraltro anche nella risposta, agli uffici giudiziari di Bari. Resta peraltro, soltanto in termini di impegno e quindi in termini di ipotetica prospettiva futura, una risposta molto labile in ordine alla gravità, denunziata dagli uffici della procura e comunque già portata a conoscenza dal sottoscritto nella passata legislatura con analoghi atti di sindacato ispettivo, della situazione relativa all'inadeguatezza degli organici. Né d'altra parte si può considerare felice la situazione degli uffici giudiziari di Bari, in ragione del fatto che si trovano in una condizione meno peggiore di quella di altri uffici giudiziari del nostro Paese; nostro Paese; resta una situazione particolarmente grave e critica, in considerazione non soltanto del *deficit* di organico. Si pensi che, soltanto nel corrente anno, soltanto nel corrente anno, ben dieci impiegati raggiungeranno l'età prossima al pensionamento ed è noto che il bando di mobilità per ora prevede l'assegnazione di una sola unità di personale. Attesa anche la situazione di particolare gravità denunziata dagli uffici della procura per l'area distrettuale di Bari per quanto attiene alla complessità e alla virulenza degli atti criminosi compiuti dai *clan* mafiosi operanti nel territorio di Bari, ma anche di Foggia (si pensi che, negli ultimi anni, sono stati registrati oltre 200 omicidi mafiosi, senza parlare della lunga striscia di sangue, che si allunga fin dietro la porta delle istituzioni),

viene anche denunciata l'assoluta insufficienza delle iniziative legislative poste all'attenzione del Parlamento dal Governo, licenziate dallo stesso Parlamento, che avevano una tendenza deflattiva e che invece, viene evidenziato, addirittura hanno un effetto di ulteriore aggravio delle incombenze e duole constatare che non si prevede alcun tipo di di integrazione o modifica alle vigenti norme, anche le più recenti, approvate dal Parlamento con la finalità di avere un effetto deflattivo sul sistema.

con l'atto ispettivo in esame, l'onorevole interrogante affronta una serie di questioni attinenti all'esecuzione della pena ed al sistema penitenziario, con specifico riferimento alla casa circondariale di Taranto e ad un episodio di rivolta dei detenuti ivi occorso. Dalla relazione trasmessa dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria risulta che, effettivamente, il 30 aprile 2016, presso la sezione B dell'istituto penitenziario di Taranto, si è verificata una protesta collettiva dei detenuti, nel corso della quale un agente della polizia penitenziaria ha subito una violenta aggressione. La stessa, tuttavia, è stata tempestivamente ed efficacemente contenuta ed i detenuti individuati come promotori sono stati sanzionati disciplinarmente e trasferiti per ragioni di sicurezza in altre sedi penitenziarie al di fuori della Regione. Con specifico riguardo alle risorse umane assegnate alla casa circondariale di Taranto, deve rilevarsi che risultano attualmente in servizio 293 unità di personale di polizia penitenziaria e che la scopertura rispetto alla previsione organica è di 46 unità, per cento del totale, pressoché in linea con il dato nazionale. Per fronteggiare la scopertura, nel corso del 2015, è stato assegnato al personale del carcere tarantino tarantino un monte ore di straordinario di 65.050 ore (che corrispondono ad un apporto lavorativo di circa 30 unità di personale al giorno), che non è stato necessario impiegare per intero, essendone state utilizzate 63.396. In linea generale, il Ministero riserva particolare attenzione alle condizioni di lavoro del personale di polizia penitenziaria, al quale è stato dedicato anche uno specifico tavolo tematico nell'ambito degli Stati generali sull'esecuzione penale, iniziativa da poco conclusa. Al fine di adeguare l'organico del Corpo di polizia penitenziaria alle esigenze organizzative ed alle finalità trattamentali, già nel 2014 il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ampliato la dotazione di risorse umane fino a 45.325 unità e - con la legge di stabilità per l'anno in corso, grazie all'impegno profuso da questo Ministero, sono state stanziate le risorse economiche necessarie per procedere al riallineamento dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con quelli corrispondenti delle altre forze di polizia. La concreta realizzazione di tale previsione è demandata ad un provvedimento normativo, per la cui elaborazione è attualmente in corso un'analisi congiunta con il Ministero dell'interno, nell'ambito del riordino complessivo delle forze di polizia. Analogo impegno viene profuso sul fronte del miglioramento delle strutture penitenziarie. Deve, al riguardo, farsi riferimento ai lavori del tavolo paritetico, istituito tra il Ministero della giustizia ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione di importanti interventi volti al miglioramento delle condizioni di vita, tanto del personale quanto dei detenuti, attraverso un piano di ammodernamento delle strutture penitenziarie in grado di allinearle agli *standard* previsti a livello europeo, secondo il Piano carceri oggetto di continua verifica ed aggiornamento. Le iniziative citate hanno interessato anche la Regione Puglia attraverso la realizzazione di importanti interventi, in corso di esecuzione presso le strutture di Lecce e Taranto. In particolare, per l'istituto penitenziario tarantino sono stati già da tempo avviati i lavori di recupero strutturale del blocco C e del reparto osservazione. Specifici interventi hanno recentemente riguardato, inoltre, gli spazi comuni, destinati alle attività sociali ed al culto, nonché le aree verdi destinate alle attività trattamentali e ricreative ed ai colloqui con i figli minori. Sono già stanziate, inoltre, le risorse per consistenti ristrutturazioni presso le case circondariali di Brindisi, Bari e Trani. Grazie a tali iniziative, la capienza detentiva della Regione Puglia - che attualmente dispone di 2.359 posti - sarà ulteriormente incrementata di 600 posti. Con riguardo poi all'ulteriore quesito sollevato dall'onorevole interrogante - con il quale viene espressa preoccupazione in merito al rischio di intimidazione degli operatori penitenziari - deve essere evidenziato che all'interno degli istituti penitenziari viene operato un costante e capillare monitoraggio, realizzato in stretta collaborazione con le procure della Repubblica territorialmente competenti. Per quanto concerne, infine, la complessa questione della transizione dagli ospedali psichiatrici giudiziari alle REMS, va preliminarmente precisato che la competenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è stata circoscritta a seguito dell'accordo sancito nella Conferenza unificata il 26 febbraio 2015, ed è limitata a fornire all'autorità giudiziaria l'indicazione della struttura residenziale di riferimento per il ricovero delle persone raggiunte dal provvedimento applicativo della misura di sicurezza detentiva. Ricade, invece, nella competenza del Ministero della salute e dell'amministrazione regionale la materiale esecuzione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria. Come noto, la mancata realizzazione da parte delle Regioni di un numero di posti letto sufficiente ad accogliere le persone sottoposte alle misure di sicurezza detentive ha determinato una situazione di generale criticità. Tale situazione, tuttavia, è in corso di risoluzione, a seguito del commissariamento delle Regioni inadempienti disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ottobre del 2015 ed alla nomina, nello scorso febbraio, del commissario straordinario, recentemente rinnovata per ulteriori sei mesi. Grazie ai significativi sforzi compiuti anche dalla Regione Puglia, sono state infatti attivate le REMS di Spinazzola e di Carovigno che offrono, rispettivamente, 20 e 18 posti, in linea con quanto stabilito con la programmazione generale presentata ed approvata per il finanziamento dallo stesso Ministero. Più in particolare, la REMS di Spinazzola, dotata di 20 posti letto, è entrata in funzione il 25 novembre 2015 ed ha raggiunto in breve tempo la capienza recettiva massima. Con la recente attivazione della REMS provvisoria di Carovigno si è, infine, potuto dar corso ai trasferimenti degli internati della Regione Puglia già ospitati presso gli ospedali psichiatrici giudiziari di Barcellona Pozzo di Gotto e di Caltagirone. La questione della limitata capienza delle strutture è affrontata anche nell'ambito dell'Atto Senato 2067, recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena», attualmente in discussione al Senato. Il Governo presterà particolare attenzione a tutti gli spunti di riflessione ed alle soluzioni che potranno emergere dal dibattito parlamentare. Nella prospettiva di assicurare il più adeguato trattamento terapeutico ai detenuti affetti da infermità psichica sopravvenuta nel corso della restrizione, è stata anche prevista presso la casa circondariale di Lecce l'attivazione di una sezione denominata «Articolazione per la tutela della salute mentale», realizzata con criteri tali da permettere l'espletamento degli accertamenti di cui all'articolo 112 del decreto I lavori per l'adeguamento della sezione sono stati ultimati e, per la sua effettiva attivazione, si attende che la ASL di Lecce ultimi le procedure di competenza del servizio sanitario regionale. Quanto sin qui riferito dimostra l'attenzione che le politiche del Ministero della giustizia riservano a tutte le questioni legate all'esecuzione della pena e si rassicura l'onorevole interrogante sull'impegno che il Governo continuerà a dedicare a questo cruciale settore.

Visito da circa dieci anni i penitenziari della mia Regione e devo evidenziare che, per quanto riguarda in particolare il penitenziario di Taranto, a fronte di un organico previsto di 340 unità,

che i dipendenti e, particolarmente, gli organi di polizia penitenziaria svolgono unitamente ai ruoli amministrativi e direzionali nell'esercizio delle loro funzioni. In più, si consideri delle 288 persone in servizio a Taranto, 118 sono con età superiore a cinquant'anni e 145 hanno più di venticinque anni di servizio e 58 godono delle agevolazioni

sovraccarico per un lavoro che di per sé è particolarmente usurante. Non trovo inoltre soddisfacente la risposta in relazione all'impegno assunto dal Governo sul versante della realizzazione delle REMS. È vero che abbiamo avuto in Puglia l'attivazione di due REMS, una a Carovigno e una a Spinazzola, però informo il Sottosegretario che, con l'interrogazione presentata in data odierna, interrogo il Ministro della giustizia in ordine ad una patologia gravissima, della quale vorrei si prendesse carico sin d'ora, relativa all'illegittima detenzione di una detenuta presso il penitenziario di Taranto, la quale dovrebbe essere invece inviata in una REMS

a Spinazzola la predetta detenuta, si è riscontrato il diniego all'ospitalità per carenza di posti e, quindi, questa persona che, per ordine del gip, deve essere detenuta in una REMS, oggi è illegittimamente detenuta presso il carcere di Taranto. Credo si tratti di una patologia particolarmente grave dal punto di vista dell'organizzazione del sistema che naturalmente impone interventi efficaci che, spero, possano essere realizzati, ma che non mi pare nella nota di risposta vengano indicati come immediati nell'imminente prossimità.

gli onorevoli interroganti paventano - nel contesto di una più ampia ricostruzione degli esiti della revisione delle circoscrizioni giudiziarie - la soppressione di alcuni uffici giudiziari sardi, con sacrificio del principio di prossimità della giurisdizione, secondo le conclusioni rassegnate dalla commissione ministeriale per la riforma dell'ordinamento giudiziario. Chiede, pertanto, se e in che termini il Ministro intenda attuare le linee riformatrici tracciate nella relazione conclusiva dei lavori. Come noto, il Ministero della giustizia ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012, e successive modificazioni. La revisione dei tribunali ordinari ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione. La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa. Il processo di revisione della geografia giudiziaria è pertanto sottoposto a una verifica progressiva ed è ulteriormente orientato alla ridefinizione degli uffici di secondo grado. Con riferimento agli uffici distrettuali, infatti, l'analisi dei dati statistici evidenzia che la distribuzione dei carichi di lavoro presso le singole corti di appello è estremamente eterogenea sia per il settore civile, che per il settore penale, con disequilibrata distribuzione degli affari tra gli uffici. Si è imposta, pertanto, l'esigenza di nuovi interventi in materia di geografia giudiziaria, con specifico riferimento all'assetto degli uffici di secondo grado. Il Ministro ha pertanto istituito una commissione di studio, presieduta dal professor avvocato Michele Vietti, a cui sono state demandate attività di analisi e di studio finalizzate alla formulazione di proposte normative, nella generale prospettiva dell'aggiornamento e della razionalizzazione del sistema secondo i principi dettati dalla Carta costituzionale e con l'obiettivo dell'efficienza nella resa di giustizia, anche con specifico riferimento allo sviluppo del processo di revisione della geografia giudiziaria. In questa prospettiva, la Commissione ha elaborato un intervento che si propone di portare a compimento il processo di razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, finalizzato ad incrementare anche l'efficacia degli uffici di secondo grado e a realizzare risparmi di spesa pubblica, attraverso la ridefinizione dell'assetto territoriale dei distretti delle corti di appello, anche mediante l'attribuzione di circondari di tribunali appartenenti a distretti limitrofi, secondo i criteri oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze. Oltre che di tali criteri, e nella prospettiva indicata dall'onorevole interrogante - lo studio della commissione ha considerato la specificità territoriale del bacino di utenza, inclusa la peculiare situazione infrastrutturale, nonché la misura dell'impatto del riassetto degli uffici sulle esigenze di contrasto dei fenomeni criminali come connotati nei singoli territori di riferimento, nella ricerca di un bilanciamento tra i vari interessi coinvolti che consenta di individuare le soluzioni più adatte a migliorare l'efficienza della giustizia al servizio del cittadino. Nella prospettiva di assicurare il più ampio confronto istituzionale e di acquisire ulteriori elementi di riflessione, la commissione ha svolto anche opportune interlocuzioni con il Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio nazionale forense, l'Associazione nazionale dei magistrati. All'esito dei lavori e tenuto conto del fatto che le proposte formulate si offrono al più ampio dibattito politico e istituzionale, ulteriori valutazioni potranno essere sottoposte all'esame del Governo per l'avvio del percorso parlamentare delle opportune iniziative normative. Il contenuto tecnico dei progetti normativi che prenderanno progressivamente forma dovrà pertanto essere ancora delineato e più ampiamente discusso. Le proposte formulate saranno, allo stato, suscettibili di ulteriori riflessioni e valutazioni, soprattutto in riferimento a specifiche realtà territoriali.

in relazione all'atto ispettivo con cui gli onorevoli interroganti chiedono di sapere se alla dottoressa Silvana Saguto, già presidente della prima sezione penale e per le misure di prevenzione del tribunale di Palermo, sia ancora assegnato il servizio di tutela, deve essere preliminarmente precisato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6

la procedura di assegnazione delle misure di tutela e protezione nei confronti delle alte personalità istituzionali, nonché delle persone che, per le funzioni esercitate o per altri comprovati motivi, sono soggetti a pericolo o minacce, è assegnata alla competenza del Ministero dell'interno e, più in particolare, all'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale. Secondo la citata normativa, ricade, altresì, nella competenza del predetto Ministero dell'interno anche l'adozione dei dispositivi tutori nei confronti dei magistrati, oltre alla gestione del personale impiegato nel servizio di tutela. Nel merito della specifica vicenda oggetto dell'atto ispettivo, la prefettura di Palermo ha comunicato che il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in data 11 maggio 2016, aveva disposto nei confronti della dottoressa Silvana Saguto la misura di sicurezza della «tutela su auto specializzata» (tutela III livello di rischio), nella sua configurazione ordinaria, con esclusione del rafforzamento già disposto in suo favore dal 2013, integrata da un sistema di vigilanza generica radio-collegato all'abitazione, e con validità fino al 31 agosto 2016, salvo ulteriore verifica. Con nota in data 14 settembre 2016, il Ministero dell'interno ha comunicato che, nel quadro della periodica revisione delle misure di protezione, la riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia presso la prefettura di Palermo ha riesaminato il grado di esposizione a rischio della dottoressa Saguto e, su proposta del prefetto, l'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale del dipartimento della pubblica sicurezza ha attenuato la misura di protezione personale, portandola portandola dal terzo al quarto livello di rischio, così adeguandola alle attuali esigenze. Preme ribadire che si tratta di misure di tutela che vengono adottate dalla competente autorità di pubblica sicurezza.

però ci sono molti soggetti che vengono tenuti sotto scorta anche quando il pericolo è venuto a mancare. Molte volte, queste scorte, quando arrivano al quarto livello, essere dei semplici accompagnatori. Sappiamo tutti che è molto difficile arrivare alla revoca della scorta, anche quando in realtà

della sezione delle misure cautelari del tribunale di Palermo, ed è stata prorogata un'inchiesta per corruzione, induzione e abuso di ufficio. Si tratta di fatti molto gravi perché la procura di Caltanissetta sta ancora indagando sugli illeciti nella gestione dei beni sequestrati a cosa nostra, che coinvolge oltre alla dottoressa Saguto anche alcuni dei suoi familiari, amministratori e magistrati, e la proroga serve proprio per continuare ad indagare su una quarantina di amministrazione giudiziarie. Da quando ho presentato l'interrogazione, devo dire che si è esteso questo cerchio magico, fatto di favori e regalie nelle amministrazioni, di ricchezze sottratte ai *boss*, creando un sistema che viene descritto come la mafia dell'antimafia.

beni sequestrati con l'antimafia, sia ancora considerato a rischio e venga tenuto sotto scorta.